Grazie

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della difesa, il Ministro dell'istruzione e il Ministro per gli affari europei. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso, ovvero tre minuti per l'interrogante, tre minuti per il Ministro e due minuti per la replica.

dovrà essere ancora più efficace per superare la vergognosa, costante e continua campagna dei *no vax* contro tale strumento. Stiamo vivendo un periodo in cui abbiamo già sperimentato, signor Ministro, la

realizzare l'immunità di gregge e, per fare ciò, signor Ministro, abbiamo bisogno di vaccinare almeno 40 milioni di italiani. E tutto questo dovremo farlo in pochissimo tempo. È solo con l'immunità di gregge che siamo riusciti, negli anni, a sconfiggere la poliomielite, il vaiolo e altre malattie. Ed è solo con l'immunità di gregge che riusciremo a garantire tutte le persone che non potranno vaccinarsi, perché sottoposte a chemioterapia e, quindi, immunodepresse. Questo è ciò che dobbiamo spiegare costantemente. La vaccinazione di massa serve innanzitutto a quelle persone. Naturalmente, per fare tutto questo, per vaccinare 40 milioni di italiani, almeno, in poche settimane, c'è bisogno di un impegno straordinario e non possiamo affidarci soltanto a coloro cui ci siamo affidati per la vaccinazione antinfluenzale:

nonché per la distribuzione e la somministrazione del vaccino. Non le chiediamo se siete pronti, perché l'Esercito è pronto per definizione. Non le chiediamo l'impegno, perché ci fidiamo del suo impegno, signor Ministro. Le chiediamo cosa state facendo materialmente per

ribadire che, sin dai primi giorni dell'insorgere dell'emergenza, le Forze armate hanno fornito il loro apporto, esprimendo capacità diversificate che sono state messe - e sono - a disposizione della collettività, e continueranno a farlo, rispondendo alle necessità e ai bisogni del Paese con una presenza continua e costante al servizio dei cittadini. Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, il personale militare, sanitario e non,

per il lavoro che, senza sosta, svolgono dall'inizio della pandemia. *(Applausi)*. Attualmente sono impegnati, tra gli altri, 1400 militari per l'operatività di 200 *drive through*, in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno. A ciò vanno aggiunti il quotidiano lavoro e l'impegno del personale impiegato nei laboratori diagnostici a Taranto e Ancona, negli ospedali da campo e presso gli ospedali militari di Milano e del Celio. Nell'attuale fase emergenziale, per quel che riguarda il tema posto dell'interrogante, la guida e il coordinamento del processo finalizzato alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19, sono in capo al Ministero della salute, per quel che riguarda la definizione del piano strategico, e del commissario straordinario, dottor Domenico Arcuri, per la definizione degli aspetti logistici organizzativi, in particolare relativi ai processi di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini, fondamentali per la realizzazione del piano strategico stesso. La Difesa partecipa, fin dalla sua costituzione, al gruppo di lavoro intersettoriale del Ministero della salute sui vaccini e vaccinazioni anti Covid-19, istituito con decreto direttoriale del 4 novembre 2020, e lavora stabilmente con il commissario straordinario che - per esempio - proprio questa mattina sta incontrando il comandante del Comando operativo interforze, sotto la cui direzione ricadono tutte le missioni della Difesa, tra cui anche quelle relative all'emergenza sanitaria in corso. In tale quadro di coordinamento, la Difesa - come ha sempre fatto dall'inizio della pandemia - fornisce e fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità predisposte in termini di concorso delle Forze armate alla distribuzione e alla somministrazione del vaccino alla popolazione italiana. In tale ottica, il Comando operativo interforze ha già avviato il processo di pianificazione, che prevedrà - per quel che riguarda il contributo alla distribuzione del vaccino - l'impiego, se ritenuto necessario dalle suddette autorità, delle infrastrutture logistiche e degli assetti di trasporto delle Forze armate; per quanto riguarda la somministrazione, l'ampliamento e la trasformazione della rete dei *drive through* presenti in tutto il territorio; infine, per eventuali esigenze specifiche, quali - per esempio - l'intervento presso i presidi residenziali per anziani, la composizione di *team* sanitari mobili pronti all'occorrenza. La Difesa quindi è pronta a rispondere con tutte le sue risorse di personale, mezzi e strutture alle esigenze che saranno rappresentate dalle autorità competenti, come ha fatto con professionalità e dedizione sin dall'inizio dell'emergenza pandemica.

Non avevo dubbi sul fatto che vi fossero, da parte delle Forze armate del nostro Paese, una disponibilità e un'organizzazione adatte ad affrontare una sfida che fa tremare i polsi, perché vaccinare milioni di italiani in poche settimane non sarà per nulla semplice. Bisognerà farlo in luoghi non affollati, per evitare ulteriori contagi; ci sarà poi bisogno di un secondo richiamo. Quindi, la mobilitazione sarà enorme e il vostro ruolo sarà indispensabile. Sono pertanto soddisfatto della sua risposta. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo a chi

- Premesso che: in considerazione dell'attuale scenario nazionale ed internazionale, nonché della rilevanza geopolitica e geostrategica acquisita dalla dimensione cibernetica

mondiale abbia aumentato gli scenari di crisi ed accresciuto i fronti di vulnerabilità e di permeabilità dei sistemi di sicurezza nazionali, mentre si registra contestualmente crescente preoccupazione in ordine all'*escalation* della minaccia terroristica internazionale, anche purtroppo alla luce dei più recenti attentati. Pertanto, ogni questione relativa al potenziamento di tutte le attività di *intelligence* rappresenta una scelta organizzativa e strategica di preminente interesse nazionale. In tale contesto resta purtroppo ancora in stallo, tra gli Stati membri, l'Accordo sul bilancio 2021-2027 nella Next generation EU, cruciale anche nel settore della difesa e della sicurezza, a cominciare dal cosiddetto Fondo europeo per la difesa. Il Consiglio dell'Unione europea del 20 novembre scorso, che si è svolto in videoconferenza - quello, per intenderci, interrotto con un atto di pirateria informatica da un giornalista francese - ha approvato 47 progetti, compresi quelli del settore della *cyber* difesa, ed ha avviato, con la condivisione dei primi documenti di *intelligence*, il processo di elaborazione dello *strategic compass*, cioè un documento

alla *cyber security* e alla *cyber defence*. Si chiede quindi di sapere, Ministro, quali siano le iniziative di competenza che si intende adottare in tema di difesa e sicurezza cibernetica per la tutela degli interessi nazionali, nonché quale sia il coinvolgimento - lo sottolineo dell'industria della difesa italiana su questo fronte di prima trincea.

dei ministri del 17 febbraio 2017. Questo decreto attribuisce al direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) l'autorità di adottare le iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione per innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, con particolare riguardo alle azioni di prevenzione, contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica. In questo contesto la Difesa prende parte attiva nelle iniziative interministeriali di attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, fornendo in particolare il proprio contributo ai lavori di definizione dei decreti attuativi del decreto-legge 21 settembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Ciò premesso, il Dicastero è dotato di assetti di cybersicurezza, inquadrati nell'ambito del neocostituito Comando per le operazioni in rete (COR), responsabile della condotta dell'operazione nel dominio cibernetico e della gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti gli assetti strategici per le telecomunicazioni, incluse quelle satellitari, per la cui realizzazione e il mantenimento in operatività sono stati effettuati significativi investimenti in termini di risorse umane e finanziarie. Tali misure sono finalizzate a esercitare le funzioni circoscritte al perimetro di operatività della Difesa, stabilito dal vigente quadro normativo, in particolare dal COM e dal Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale. In tempo di pace tali funzioni si sostanziano nella protezione delle reti e dei sistemi informativi della Difesa, nella sorveglianza sui possibili attacchi portati alla infrastruttura ICT, nel mantenimento di prontezza operativa necessario a un efficace contrasto della minaccia *cyber* e, non ultimo, nell'eventuale attività di supporto, richiesta nell'ambito del nucleo per la sicurezza cibernetica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di incidente informatico occorso a qualsivoglia infrastruttura nazionale. In ambito internazionale, inoltre - come ha ricordato l'onorevole senatrice interrogante - la Difesa è coinvolta sulle tematiche *cyber* sia nel contesto dell'Alleanza atlantica che in quello dell'Unione europea, partecipando, con fattivi contributi, a tutti i tavoli volti a incrementare la sicurezza cibernetica. Questi ambiti rappresentano importanti banchi di prova e confronto per l'innalzamento del livello nazionale e dell'Alleanza nel dominio *cyber*. Nel quadro che ho ora illustrato e nei limiti del mandato ricevuto, che non prevede l'erogazione di servizi di sicurezza a favore di aziende private italiane non solo private), il Dicastero ha delineato la programmazione degli investimenti nella dimensione digitale e, in particolare, di quelli afferenti la cybersicurezza, assegnando le priorità ai principali progetti di ammodernamento e trasformazione dello strumento militare, rispettando i princìpi di sostenibilità, delle capacità di capitalizzazione delle risorse investite e di condivisione in ambito interforze dei processi di acquisizione, e proseguendo la sinergia, da tempo avviata, nel campo della ricerca con le università e con l'industria, come da lei citato.

non sono insoddisfatta della sua risposta, ma come Fratelli d'Italia siamo e restiamo insoddisfatti per i contenuti del Documento programmatico pluriennale della difesa e soprattutto per i finanziamenti, che ci appaiono purtroppo inadeguati, come sono inadeguati gli investimenti e - com'è e - com'è a tutti noto - quel disallineamento nel *budget* nazionale della Difesa rispetto al previsto 2 per cento del PIL per i Paesi dell'Alleanza. Tuttavia, insisto proprio sull'aspetto del dominio cibernetico, che è la vera frontiera delle contese geopolitiche e atteso che competenza su questa materia

grazie a tutti è l'asse strategico per la sicurezza di ogni sistema nazionale e, quindi, anche per il nostro. Nel Documento programmatico la parola «*cyber*» appare 13 volte; la parola «*cybersecurity*» 9 volte; le parole «*cyber defence*» 8 volte; la parola «cibernetico» 33 volte e più, mentre la parola «*intelligence*» compare

camion, all'esigenza di maggiori pietà, soccorrendo i defunti in un momento in cui la prima ondata del virus sembrava mettere in ginocchio lo Stato. Da allora, in diverse occasioni le Forze armate hanno raccolto più

Le Forze armate stanno intervenendo in prima linea e, quindi, l'elogio di Forza Italia è pieno e convinto. Tuttavia, la sanità militare ha subito negli anni molti tagli. Ricordo quando, negli anni passati, in Parlamento si parlava della sanità militare come di un retaggio della Prima guerra mondiale o di epoche per fortuna lontane. Purtroppo, in altri contesti e per altre esigenze, la sanità militare si rivela importante. Aver tagliato risorse e chiuso ospedali è stato un errore. Noi di Forza Italia stiamo sostenendo il Documento della difesa perché è non un giudizio sul Governo, ma un sostegno alle Forze armate, che sono una struttura fondante dello Stato. E lo facciamo anche se siamo sotto la media che la NATO ci indica per le spese militari; lo facciamo per vicinanza alle Forze armate, all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, ai Carabinieri e a tutto il comparto della sicurezza e della difesa: penso alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, alla Polizia penitenziaria, ai Vigili del Fuoco e ad altre realtà anche della Protezione civile. civile. Noi chiediamo che vengano stanziate più risorse per la sanità militare, che non può essere invocata nell'urgenza. Ogni giorno un sindaco o un Presidente di Regione chiede l'ospedale da campo e l'intervento delle Forze armate, che agiscono; ma, se fossero state supportate meglio e di più nel tempo, potrebbero in maniera più adeguata, e senza sacrifici enormi. In questo contesto, signor Ministro, le ricordo il personale delle Forze armate, a favore del quale occorrono meno pacche sulle spalle e più risorse. Ci sono contratti da rinnovare, indennità da verificare e straordinari da compensare. Il Governo non ha nemmeno fatto l'incontro che la legge prescrive alla vigilia della manovra di bilancio. L'ultimo risale ai Governi Berlusconi, e poi non vi sono più stati. Signor Presidente, le chiediamo - la Commissione difesa del Senato lo ha chiesto con un voto unanime - che il Governo incontri tutto il comparto. A lei compete il COCER, ma il Governo, nella sua collegialità, deve estendere questo incontro ai sindacati delle altre Forze di polizia e del soccorso pubblico. Con questa interrogazione chiediamo pertanto sostegno alla sanità militare, ma attraverso fatti, per quello che noi chiamiamo il popolo in divisa.

mi sia consentito ricordare come fin dall'esordio della crisi la Difesa ha garantito la disponibilità di strutture militari per la sorveglianza sanitaria e ha messo a disposizione centinaia di medici e infermieri militari; ha inoltre fornito un robusto sostegno logistico, contribuito a garantire il controllo del territorio, l'allestimento di ospedali da campo, l'effettuazione di trasporti terrestri e aerei, invio e contenimento. Sono stati conseguiti in tempi rapidissimi il potenziamento dei centri ospedalieri di Taranto e Milano e l'adeguamento capacitivo del Policlinico militare del Celio a Roma, realizzando un Covid *hospital* che costituisce un importante centro di riferimento per l'emergenza sanitaria nel Centro Italia, nel quadro di una rete nazionale di strutture dedicate al contrasto della malattia. Significativo è anche il sostegno fornito alle aziende del settore sanitario, che ha permesso ad alcune di esse di moltiplicare la produzione, contribuendo al raggiungimento dell'autonomia nazionale per la realizzazione di presidi medici essenziali. Più di recente, in relazione all'attuale recrudescenza del contagio, è stata fornita la disponibilità di assetti della sanità militare per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi attraverso l'avvio dell'operazione Igea. Il personale sanitario militare ammonta a circa 3.810 unità, di cui 1.185 ufficiali medici, 56 farmacisti, 95 veterinari, 154 psicologi, 32 odontoiatri, 8 biologi, 1.833 sottufficiali delle professioni sanitarie (infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici ortopedici, audiometristi, igienisti dentali) e ulteriori 147 medici e 300 infermieri arruolati per le esigenze Covid con ferma per un anno. A ciò vanno aggiunti 1.493 operatori sanitari non specializzati. Nonostante negli ultimi quindici anni si sia verificata una sensibile contrazione delle risorse del bilancio della Difesa, che evidentemente ha coinvolto anche la componente sanitaria, negli ultimi quattro anni sono stati destinati al potenziamento della sanità militare oltre 85 milioni di euro, cui si aggiungono 150 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2020-2021 recati dai recenti provvedimenti emergenziali cura Italia e rilancio: una scelta ha consentito la realizzazione delle potenziate e diversificate capacità mediche e di logistica sanitaria prontamente messe a disposizione e a supporto del Servizio sanitario nazionale e dell'intero sistema Paese. In quest'ottica, come Ministro della difesa intendo confermare e rinnovare la disponibilità totale delle Forze armate nell'attuale periodo di crisi, che potrà essere ulteriormente riarticolata e potenziata, qualora ritenuto necessario, con ulteriori investimenti mirati al progressivo incremento del personale sanitario specialistico già in atto con i recenti annullamenti proposti dal Governo.

ho avuto modo di rappresentare come le difficoltà incontrate nella costruzione della complessa legge di bilancio in questa fase emergenziale non avessero favorito questo preventivo confronto, esprimendo al contempo l'impegno di portare la tematica all'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri, che mi ha già assicurato piena disponibilità a procedere in questo senso.

l'impegno all'ascolto del comparto sicurezza e difesa che lei ci ha ribadito giorni fa anche in Commissione, qui in Senato, dove - ripeto - l'unanimità dei colleghi chiede il rispetto delle leggi di ascolto del comparto. Capisco gli impegni del Presidente del Consiglio,

colleghi, sugli 800 milioni per i parlamentari. Non sono soldi che si danno i parlamentari, ma solo soldi lasciati dalla legge di stabilità per la copertura dei numerosi emendamenti che il Parlamento propone. Questo va chiarito. Il nostro Gruppo chiederà, però, che quegli 800 milioni possano essere indirizzati al comparto sicurezza e difesa: ci saranno emendamenti parlamentari in materia, e ho appena citato quello di Forza Italia; usiamo il fondo destinato alle scelte del Parlamento grazie a tutti gratitudine al popolo in divisa, in particolare alla sanità militare, che agisce anche in ristrettezza di mezzi. Grazie al popolo in divisa.

pongo una questione che in questo momento potrebbe sembrare marginale, ma credo che il tema delle istituzioni educative, dei convitti e del loro personale educativo rappresenti comunque un tassello importante per A quanto risulta, oggi non è ancora stato bandito il concorso nazionale per personale educativo e l'ultimo - di cui ho qui il bando - è stato fatto nel 2000, e poi non c'è stato più nulla. Considerato che i posti vacanti, per quanto riguarda il personale educativo, sono in continua crescita e destinati ad aumentare, a seguito del raggiungimento dei requisiti di pensionamento, che il precariato comporta a livello sia scolastico sia personale sono del tutto logoranti. Faccio un esempio: anche in Valle D'Aosta, come in altre Regioni, in seguito anche a una segnalazione di rappresentanti sindacali, si sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia relativamente alla reperibilità del personale educativo. per fare un esempio, presso l'istituzione scolastica "Convitto regionale F. Chabod" della Valle d'Aosta, il numero di posti attualmente vacanti e messi a supplenza come educatore è assai rilevante;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda procedere al reclutamento del personale, attraverso la pubblicazione del bando di concorso nazionale per il personale educativo, eventualmente specificando entro quali termini. **Interrogazione

senatore Laniece ben sa, i convitti e gli educandati concorrono al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano, sia tramite l'offerta formativa delle scuole a cui sono ammessi sia con i fondamentali servizi resi dalle strutture residenziali e semiresidenziali. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati della Repubblica n. 81 del 2009. Per l'anno scolastico in corso, la dotazione organica è pari a 2.279 unità. Posso assicurarle che, anche in questa difficile congiuntura, abbiamo lavorato per disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo in tempi congrui, proprio per garantire stabilità ai ragazzi, che si avvalgono del servizio dei convitti e degli educandati. Per l'anno scolastico 2020-2021 è stata autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di 91 unità di personale educativo. Venendo al quesito, è evidente che il contesto sociale in cui sono nati tali istituti è fortemente cambiato. Il numero di convittori e semiconvittori, infatti, ha registrato nel corso degli anni una contrazione, che ha conseguentemente portato ad un esubero del personale educativo di ruolo. In ogni caso tale esubero nazionale non ha comportato l'impossibilità di intervenire con le assunzioni necessarie. Sono state utilizzate, ove necessario, le graduatorie capienti ancora vigenti. Posso rassicurare l'interrogante che, al pari di tutte le altre categorie di personale scolastico, la programmazione di un fabbisogno di assunzioni si accompagnerà alle necessarie procedure concorsuali, secondo quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione. Preciso solo, con riferimento alla richiesta riguardante la Regione autonoma Valle d'Aosta, che i concorsi per il reclutamento di detto personale sono indetti dalla Regione stessa in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi banditi nel restante territorio nazionale. Nondimeno assicuro ogni contributo mio e della struttura che rappresento che possa fornire, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un utile e qualificato apporto per la valorizzazione e il rilancio di tali istituzioni che costituiscono indubbiamente un patrimonio della nostra comunità.

urge un cambio di passo affinché nell'attuale crisi economica, occupazionale e sociale diventino davvero prioritarie la questione educativa e l'effettiva pluralità dell'offerta scolastica. A tal fine si ritiene necessario prendere in considerazione quattro possibilità: la sottoscrizione di patti educativi di comunità, che coinvolgano il Ministero dell'istruzione, le Regioni e i Comuni, generando un'alleanza tra le 40.000 scuole statali e le 12.000 paritarie, al fine di reperire locali e mezzo di trasporto che consentano a tutti di frequentare, alle stesse condizioni, una statale o una paritaria, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà per la pandemia o che condividono l'esperienza della disabilità; prevedere un incremento di risorse per il pluralismo scolastico in riferimento alla qualità e alla continuità del servizio offerto dalle paritarie, di cui alla legge n. 62 del 10 marzo 2000 e, a e, a partire dall'esercizio fiscale 2021, la deducibilità della retta versata fino a 5.500 euro ad alunno; eliminare ogni discriminazione fra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria, per superare l'impari accessibilità in tema di erogazione di fondi, dotazioni e risorse, specialmente se legate alle criticità e agli oneri determinati dalla pandemia; l'incremento del fondo, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle paritarie che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo disabile la disponibilità del docente di sostegno e non imporne il costo alla famiglia o alle scuole paritarie che, chiaramente, non sono in grado di sostenerlo. Considerato che: le scuole paritarie offrono assoluta disponibilità alla rendicontazione dei contributi, rivedendo le linee di finanziamento del sistema scolastico attraverso l'introduzione dei costi standard di sostenibilità, da declinare in convenzioni, *voucher*, buono scuola, detraibilità delle rette, devoluzione del 10 per mille (misura peraltro già proposta dalla Lega con specifico disegno di legge presentato in Senato); considerato altresì che nella fase 2 del Covid-19 la scuola statale, il cui costo annuale a carico della collettività per alunno è pari a 8.500 euro, non è riuscita ad assicurare la ripartenza della didattica per tutti, mentre le scuole paritarie sopravvissute alla carenza di risorse generata dalla pandemia, con rette che vanno dai 3.800 euro per la scuola dell'infanzia ai 5.000 euro per il liceo, hanno comunque assicurato il servizio, si chiede di sapere se il Ministro intenda avviare una sinergica collaborazione, ed eventualmente in che termini, tra scuole pubbliche statali e scuole paritarie al fine di innalzare il livello qualitativo del sistema scolastico nel suo insieme, rendendolo più equo e generando, a fronte di un servizio migliore, un probabile significativo risparmio di risorse pubbliche.

e non potrebbe essere altrimenti in quanto, come noto, le scuole paritarie formano insieme alle scuole statali il sistema nazionale d'istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000. La sinergia non si esaurisce in tale collaborazione ma già coinvolge, tramite i patti di comunità da lei richiamati, enti e amministrazioni locali, nonché le realtà associative. In tal senso, determinante è stato l'investimento dei mesi scorsi finalizzato a sostenere la realizzazione, all'interno delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, proprio dei patti di comunità; accordi già fatti, che hanno stimolato e generato iniziative e buone pratiche di cooperazione che potranno essere incentivate ancor di più e promosse. Con riferimento al finanziamento per il segmento delle scuole paritarie assicurato nel corso del tempo, le evidenzio come il Ministero dell'istruzione abbia già garantito l'emanazione di tutti gli atti di propria competenza nel rispetto della legislazione vigente. Nell'ottica dell'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e formazione nel disegno di legge di bilancio, ora all'esame del Parlamento, è stato altresì previsto lo stanziamento di 60 milioni di euro a regime, a decorrere dal prossimo anno, del fondo destinato al sostegno del sistema integrato da zero a sei anni. Quanto alla previsione della detrazione Irpef delle rette e delle spese relative alla frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, ricordo che già esiste nella misura del 19 Ulteriore attenzione è stata riservata nell'emergenza. Proprio perché coscienti del ruolo delle criticità e degli oneri legati alla pandemia rispetto a tutte le istituzioni scolastiche, come da lei evidenziato, già con il decreto-legge n. 18 del marzo scorso e con il cosiddetto decreto-legge rilancio abbiamo assegnato specifiche risorse alle scuole paritarie, anche per dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e di igiene, sia per il personale che per gli studenti, oltre che per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato. Senatore, quanto fin qui illustrato dimostra che stiamo lavorando alacremente nell'interesse esclusivo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti all'interno di una cornice unitaria quella del sistema di istruzione e formazione - delineata dalla nostra Costituzione. Presidente, colleghi, non posso certo ritenermi soddisfatta della risposta. Signor Ministro, lei ha ripetuto la litania che da mesi continuiamo a sentire, ma soprattutto, lei continua a pensare che il pubblico, lo Stato, possa fare tutto da solo, e che ciò che nasce ed esiste grazie all'iniziativa privata sia solo un fardello da sostenere, mentre spesso è vero il contrario. Nell'interrogazione che abbiamo presentato le abbiamo suggerito noi stessi le parole che avremmo voluto sentire da lei, Ministro, ma lei, concentrata ideologicamente sul centralismo, anziché su quella forma di autonomia che tanto

si possono trovare le soluzioni giuste ai tanti problemi che da solo il pubblico non è in grado di risolvere, nella scuola così come in tanti altri ambiti, per esempio, nei trasporti, come apparso evidente in quest'ultimo periodo. non è un ambito di sua competenza, ma se fin da subito aveste ascoltato le proposte della Lega, mettendo in atto una collaborazione tra trasporto pubblico e privato, forse tanti studenti delle scuole superiori non sarebbero obbligati a seguire le lezioni da casa, Ministro: stessa identica cosa per quanto riguarda la scuola. La invito, Ministro, a riflettere sul fatto che è indispensabile una sinergia tra scuola statale e scuola paritaria. Solo così potremo assicurare ai nostri giovani una qualità d'istruzione eccellente, garantendo la libertà di scelta educativa e anche risparmiando risorse pubbliche. Se ancora non è convinta di questo, Ministro, mi permetta di farle solo un esempio, senza farla andare troppo lontano, ricordandole che il primo liceo STEM in Italia è stato istituito a Palermo, proprio in una scuola paritaria, che lei penso ben conoscerà. Ministro, lei sa bene di cosa stiamo parlando quando si parla di indirizzo STEM o STEAM, perché è ciò su cui si fonda il Piano nazionale scuola digitale, con l'obiettivo di innovare il sistema educativo italiano. Spero che lei faccia una riflessione su quanto le ho esposto, Ministro, e tra qualche tempo torni in quest'Aula con argomentazioni diverse; ne ha la possibilità anche a breve con la prossima

signor Ministro, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato, a partire dal mese di marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per gran parte del tempo trascorso fino ad oggi, rendendo necessario disciplinare con strumenti emergenziali dapprima le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019-2020 e, in seguito, quelle inerenti all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021. In ogni caso, nell'ambito della decretazione d'urgenza che ha riguardato il settore scolastico sono state stanziate in via progressiva risorse sempre più ingenti al fine di permettere il prosieguo delle attività in modalità digitale (didattica a distanza, didattica digitale integrata), in modo da garantire per quanto possibile la continuità didattica. Tra le misure da ultime disposte è purtroppo annoverata anche la possibilità di sospendere le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò è avvenuto in via obbligatoria in tutto il territorio nazionale per le scuole secondarie di secondo grado e per il secondo e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e sulla base di scenari di rischio articolati su base regionale per le scuole dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tuttavia è opportuno notare come uno scenario caratterizzato per la gran parte dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, fermo restando il rigoroso rispetto delle imprescindibili misure di sicurezza e prevenzione volte a contenere i contagi, possa determinare sia ripercussioni sullo stato psicologico degli studenti sia l'aumento di un fenomeno deleterio quale la dispersione scolastica, che rischia di lasciare tracce indelebili in quei contesti più degradati e caratterizzati da povertà educative e arretratezza socio-economica. Per tale ragione, la riapertura delle scuole in sicurezza si pone quale priorità assoluta nel nostro Paese. Difatti, in particolare è da sottolineare come il settore scolastico risulti particolarmente danneggiato dalle carenze afferenti tra gli altri quello dei trasporti locali. Nel panorama attuale, caratterizzato da una estrema incertezza anche nel breve periodo, è indispensabile che lo Stato investa adeguate risorse sia per la spesa corrente che per gli investimenti, in modo da garantire il più possibile il proseguo dell'attività didattica in presenza. Si chiede dunque di sapere quali misure di competenza abbia assunto il Ministro, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio in materia di scuola, sia al fine di fronteggiare in modo più adeguato l'emergenza sanitaria in corso

senatrice Granato, mai come in questo momento la scuola è tornata al centro del dibattito pubblico e mai come ora è radicata la consapevolezza che l'istruzione sia uno dei principali motori di sviluppo del nostro Paese. senatrice Granato, che stiamo investendo risorse e lavorando non solo per l'oggi ma anche per il futuro, per una scuola aperta, coesa, solidale, inclusiva e innovativa. Le significative misure previste nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, in questo momento all'esame della Camera dei deputati, ne sono un'eloquente testimonianza. È previsto un piano pluriennale per l'assunzione a tempo indeterminato di 25.000 docenti di sostegno nel cosiddetto organico di diritto, per garantire continuità didattica alle alunne e agli alunni con disabilità. Viene destinata una cifra pari a 10 milioni di euro per la formazione di tutti i docenti, non solo di sostegno, sulle tematiche inerenti all'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità. stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che li accolgono. Si è data certezza a 4.485 collaboratori scolastici ex LSU, trasformando a tempo pieno il loro contratto di lavoro, assicurando così un adeguato livello dei servizi di pulizia degli ambienti scolastici anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria. Si è anche garantita la stabilità a 1.000 assistenti tecnici per il supporto digitale nelle scuole del primo ciclo. È stata poi potenziata l'offerta formativa nella scuola dell'infanzia al fine di istituire nuove sezioni con ulteriori 1.000 insegnanti ed è stato incrementato a regime di aggiuntivi 60 milioni di euro il fondo destinato al sistema integrato da zero a sei anni. Si è investito sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (più di 100 milioni di euro nell'anno 2021), anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione soprattutto per i soggetti privi di mezzi. Allo scopo di potenziare l'innovazione didattica digitale nelle scuole sono stati inoltre investiti ulteriori 40 milioni di euro sul Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica è stato poi ulteriormente incrementato per i prossimi anni per un totale di 1,5 miliardi di euro. In totale stiamo investendo oltre 3,7 miliardi di euro. Sommando tale cifra alle risorse stanziate nei mesi scorsi, si può affermare che questo Governo ha già investito sulla scuola oltre 7 miliardi di euro. Senatrice, l'accelerazione degli investimenti, in special modo su formazione e innovazione, testimonia che in questi mesi abbiamo affrontato l'emergenza sanitaria cercando di trarne delle opportunità per il rilancio del sistema nazionale di istruzione e formazione. Sono certa che, insieme al Parlamento, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio sapremo dare ulteriori segnali di attenzione all'intera comunità scolastica.

grazie a tutti istituzionali, sia statali che territoriali, si devono quindi vedere investiti di questo importante e fondamentale impegno, perché riaprire le attività economiche senza aver prima riaperto le scuole purtroppo comporterà necessariamente che i contagi continueranno a circolare all'interno del Paese e quindi le scuole potrebbero rimanere chiuse *sine die*. Noi non possiamo permettere che una situazione di emergenza si traduca poi in macelleria sociale, perché questo sarà lo scenario dei prossimi anni se non investiamo adesso nella riapertura delle scuole. Auspico quindi che, a parte il suo impegno, vi sia anche l'impegno delle altre istituzioni per concorrere a questo fondamentale e importante obiettivo: che le scuole siano le prime ad aprire e le ultime a chiudere.

se già non bastasse il clima di sfiducia e di angoscia generati dalla pandemia in corso e dai suoi effetti sulla tenuta dei sistemi sociali ed economici dell'Italia e dell'Europa, un fatto nuovo adombra seriamente l'orizzonte e di fatto ci impedisce di agire nei tempi e nelle modalità opportune per supportare le nostre comunità in questa delicatissima fase della storia mondiale. Come sappiamo, a inizio novembre è stato raggiunto un importante accordo negoziale tra Parlamento e Consiglio dell'Unione europea sul bilancio di lungo termine e il meccanismo di ripresa, il Next generation EU, sulla base degli orientamenti politici forniti nel Consiglio europeo a luglio scorso; un accordo che ha introdotto un nuovo regime di condizionalità con l'obiettivo di tutelare ancora di più il bilancio dell'Unione europea dalle violazioni dei princìpi dello Stato di diritto. In questi giorni però stiamo assistendo ad un grave e pericoloso frangente di crisi che espone seriamente l'Unione europea al rischio di esercizio provvisorio del bilancio e, di conseguenza, ad un pericoloso ritardo nell'erogazione delle risorse destinate a risollevare l'Europa dalla profonda crisi causata dalla pandemia Covid-19. Ciò a causa dell'opposizione sollevata da Ungheria e Polonia proprio sull'inserimento del meccanismo di condizionalità che subordina l'erogazione delle risorse del bilancio europeo al rispetto dello Stato di diritto. Il veto dei due Paesi chiaramente non può essere esercitato sul meccanismo di applicazione del criterio dello Stato di diritto ai fondi europei, ma sulla decisione e sulle risorse proprie, che rischierebbe di bloccare l'approvazione all'unanimità del nuovo quadro finanziario pluriennale. Può essere utile ricordare allora non solo che l'Unione europea non è e non può essere interpretata come mero mercato economico, ma anche e soprattutto come la cornice dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali che in Ungheria e in Polonia si sta sempre più deteriorando. Giusto un giorno fa la presidente della Commissione europea ha invitato Polonia e Ungheria a rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per fugare le più che legittime preoccupazioni riguardo alla predetta condizionalità dal momento che quello è il luogo dove si disputano «i disaccordi sui testi giuridici e non a spese di milioni di europei che aspettano con urgenza il nostro aiuto». Tutto ciò è allarmante. In conclusione, signor Ministro, è per questo che le chiedo quali iniziative il Governo ritiene assumere nelle sedi istituzionali europee per garantire nei tempi necessari l'approvazione e l'immediata operatività del nuovo ciclo di bilancio, per scongiurare l'esercizio provvisorio e le gravi conseguenze che esso determinerebbe anche nell'erogazione del *recovery fund*, nonché l'introduzione del nuovo regime di condizionalità.

una questione che, come viene sottolineato, è di allarme comune e io concordo su questo allarme. L'intesa infatti del Consiglio europeo del 21 luglio scorso, quella che costruì un pacchetto da 1824,3 miliardi di euro, tra Quadro Next generation è il più ampio pacchetto di fondi finanziato dal bilancio dell'Unione europea nella storia ed è un pacchetto che è necessario per la ripresa e la resilienza e le nostre economie. Nelle conclusioni del 21 luglio scorso, ai punti 22 e 23, si scrisse quanto segue: «Gli interessi finanziari dell'Unione sono tutelati in conformità dei principi generali (...) in particolare i valori di cui all'articolo 2 TUE (Trattato

europeo e sul regolamento sulla condizionalità di bilancio che si applica appunto ai casi di violazione dello Stato di diritto. Nel negoziato con il Parlamento, le disposizioni prevedono: una funzione di protezione preventiva contro i rischi di violazione; un elenco con esempi di casi (come la minaccia all'indipendenza della magistratura); una clausola di protezione dei beneficiari finali; la possibilità di sospendere pagamenti oppure il divieto di chiedere nuovi impegni legali e anche un freno d'emergenza (vale a dire la possibilità che lo Stato membro, in violazione dello Stato di diritto, richiami la questione all'esame del Consiglio europeo). Una mediazione saggia che noi abbiamo sostenuto e questo compromesso, raggiunto nel trilogo, ovviamente deve essere adesso adottato di nuovo dal Consiglio europeo e dal Parlamento a maggioranza qualificata e, in teoria, non servirebbe il voto di Ungheria e Polonia, come lei sottolineava. In pratica, però, il veto di Budapest e Varsavia viene esercitato sul regolamento generale del QFP e sul Next Generation EU, un veto che blocca le procedure. Polonia e Ungheria motivano il loro veto riferendosi a dispute ideologiche o di violazione dei diritti. Voglio essere chiaro: si tratta di una questione giuridicamente corretta, espressa in base ai trattati e senza alcun carattere ideologico e fa bene la presidente Von der Leyen a riferirsi alla Corte di giustizia europea, perché con questo veto il pacchetto è stato bloccato l'allarme sta nel fatto che, finché questo veto non verrà superato, tutte le procedure saranno in stallo. Noi sosterremo ovviamente il ruolo della Presidenza tedesca ma permettetemi di dire che, oltre all'allarme, è una grave responsabilità...

sembra, a nome del Governo, abbia ben inteso il rischio che abbiamo di fronte. Chiedo al Ministro, a nome del Parlamento e del mio Gruppo, di tenere duro su questa linea, perché ne va della prospettiva e soprattutto questo clima di incertezza non aiuta ad affrontare ancora la crisi che abbiamo davanti e che non abbiamo risolto. Quindi la ringrazio, Ministro, di questo suo impegno e la prego di tenere il Parlamento costantemente informato, perché il clima di preoccupazione non agevola le decisioni che abbiamo davanti.

Il relatore, senatore Comincini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, già autorizzato con la precedente relazione al Parlamento allegata alla NADEF. La relazione in esame è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (la cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'obiettivo di medio termine siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentiti la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine. È opportuno ricordare che la relazione in esame è stata preceduta da quattro autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro, approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nell'anno in corso, per far fronte alla crisi economico-sanitaria da Covid-19. L'aggravamento della situazione sanitaria derivante dalla seconda ondata di contagi da Covid-19, sviluppatasi questo autunno, ha indotto il Governo ad adottare misure restrittive differenziate a livello territoriale. Le Regioni sono state suddivise in base a tre categorie di gravità delle condizioni sanitarie, a cui sono associate delle regole differenziate di distanziamento sociale e di chiusura delle attività economiche. Il quadro sanitario delle Regioni è in continua mutazione, rendendo necessario adeguare le misure di sostegno in corso di approvazione e quindi reperire risorse finanziarie aggiuntive. Chiariti i presupposti e le finalità della relazione, il Governo illustra l'aggiornamento delle stime tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso, con specifico riferimento al livello di indebitamento netto in rapporto al PIL. Nel dettaglio si rivede in miglioramento la stima dell'indebitamento netto tendenziale al 10,4 per cento del PIL, principalmente sulla scorta di una revisione al ribasso delle previsioni delle spese per consumi intermedi, redditi, investimenti e interessi. Con la relazione in esame pertanto, sentita la Commissione europea, il Governo richiede per il solo anno 2020 l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento, pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 8 miliardi in termini sia di fabbisogno sia di indebitamento netto. Per effetto della nuova richiesta di scostamento e considerando le precedenti autorizzazioni concesse e gli obiettivi programmatici definiti nella NADEF 2020 e nel documento programmatico di bilancio 2021, complessivamente il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà quindi aumentare per il 2020 fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi Per quanto riguarda il prossimo triennio di programmazione, nonostante l'elevato grado di incertezza che circonda la stima, il Governo conferma il percorso di rientro verso l'obiettivo di medio termine, già indicato nella NADEF di ottobre scorso, in base al quale

della pandemia portiamo in votazione uno scostamento di bilancio. Insisto: già per quattro volte in quest'Aula si è preso atto che il Governo sta facendo di tutto per immettere liquidità nel tessuto economico ed imprenditoriale del Paese. Siamo in un pantano, questo è chiaro, ma come dimostra questo quinto scostamento, stiamo facendo il possibile per uscirne. La situazione è costantemente tenuta sotto osservazione e si stanno adottando senza indugio le misure necessarie. D'altra parte, è innegabile che questa emergenza sanitaria mondiale è un qualcosa di mai visto nel passato. Per questo, se dovesse essere necessario, si procederà con ulteriori scostamenti per sostenere cittadini, famiglie ed imprese. Non si naviga a vista, si agisce chirurgicamente quando e dove necessario. Oggi, proprio in tale direzione, siamo chiamati a dare il via libera ad altri 8 miliardi di euro in termini di indebitamento netto: uno scostamento che forse impropriamente da qualcuno è stato definito senza *deficit*, perché sappiamo che questo importo sarà riassorbito da extra-gettito tributario, che rendiamo immediatamente utilizzabile per fronteggiare l'emergenza economico-pandemica. Chiariamo bene, per i detrattori irriducibili che non fanno altro che lamentarsi, tutti i miliardi sono stati e saranno trasferiti all'economia reale: alle piccole imprese, alla scuola, alla sanità, alle famiglie e alle partite IVA in difficoltà. Potremmo scoperchiare un vaso di Pandora per discutere di come sono stati e vengono amministrati dalle Regioni i fondi destinati all'emergenza sanitaria. Non si vuole mortificare o crocifiggere nessuno, ma dobbiamo avere l'onestà intellettuale di riconoscere che quanto stiamo purtroppo vivendo ha evidenziato in maniera inoppugnabile che una gestione centrale della sanità, di fronte a problemi così grandi, è più funzionale rispetto a decisioni regionali non unanimi. Il Titolo V della Costituzione è stato improvvidamente modificato nel passato, ma è segno di intelligenza riconoscere che bisogna rivederlo nuovamente. A tal proposito, segnalo il disegno di legge che la collega Paola Taverna ha presentato e che ho sottoscritto insieme a tanti altri. Non possiamo lasciare agli enti locali la possibilità di gestire a proprio piacimento la sanità: questo va ribadito, perché spero sia un tema centrale del nostro lavoro anche nei mesi e anni a venire di questa legislatura.

un meccanismo etichettato come superato dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli e dall'ex *premier* Enrico Letta, entrambi esponenti del PD e di una solida tradizione europeista, e da tanti esponenti di quelle stesse forze politiche che in maniera sconsiderata hanno voluto riaccendere il dibattito. Smettiamola; attingendo a quei fondi, tutt'altro che ad impatto zero, daremo un segnale devastante all'esterno. Tornando all'oggi, invece, certamente ci sono settori che sono stati toccati in maniera differente da questa crisi e che necessitano di una risposta flessibile da parte delle istituzioni.

dalla sicurezza alla ristorazione, passando per gli addetti alla posa dei materiali, la falegnameria, arredamenti per interni, il mondo della fotografia, gli appalti per le pulizie, solo per citare alcuni ambiti correlati alle fiere. Non dimentichiamo ovviamente anche tutti i quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni. Per questo, se da una parte è necessario prevedere una riapertura in sicurezza per gli enti fieristici, dall'altro abbiamo il dovere di supportare l'intero mondo fieristico svincolandoci dalla rigidità dell'impostazione dei codici Ateco. lavorare di più su tutto il mondo delle partite IVA. Lo scorso dicembre ci fu un taglio della soglia dei contratti subordinati per chi deteneva contestualmente partite IVA e regimi forfettari: una scelta miope che ha penalizzato tanti lavoratori che, in quest'anno di crisi avrebbero potuto lavorare in libera professione per arrotondare il proprio stipendio. Non si deve guardare ai professionisti e alle partite IVA come nemici da combattere. In un Paese che punta alla modernità, anche in tema di lavoro necessarie agilità e poca burocrazia, elementi che, se non perseguiti, ingabbiano il libero professionista e al contempo incentivano solamente irregolarità e abusi. Il Governo non ha mai negato la possibilità di riforme innovative per rilanciare interi settori produttivi. Il superbonus al 110 per cento, così come il bonus mobilità, sono esempi lampanti di come la politica deve incidere per risollevare il Paese, senza preconcetti e diffidenza verso i cittadini. Il superbonus al 110 per cento è un provvedimento straordinario che non potrà durare decenni, ma che sarà sicuramente prorogato coprendo un orizzonte pluriennale: un tempo congruo per avviare i cantieri in quantità, efficientando e mettendo in sicurezza le nostre case (obiettivo su cui sono certo che tutta l'Assemblea è d'accordo). La diffidenza è solo una forma di solitudine e isolamento; è quanto di più lontano ci possa essere rispetto al ruolo che ricopriamo in quest'Assemblea. Per questo motivo, credo che l'unico modo che abbiamo per rendere affidabile qualcuno sia concedergli la nostra fiducia. L'impostazione che dovremo tenere nei confronti di tutto il popolo degli imprenditori e delle partite IVA deve essere costruttivo e proattivo. Troppo spesso ho notato come il dialogo sia stato viziato da impostazioni ideologiche precostituite da una parte e dall'altra. Concludendo, plaudo all'atteggiamento di ascolto che ho trovato da parte dei Ministeri in questo periodo di difficoltà per il Paese. Le istanze hanno spesso trovato una risposta e specialmente i cosiddetti decreti ristori, in esame in Commissione bilancio in questi giorni, contengono un supporto economico a favore di moltissime categorie bloccate dai Spero che proprio con i cosiddetti decreti ristori e la legge di bilancio si possa lavorare anche con le forze di opposizione, perché siamo tutti parte di questo grande conflitto contro un nemico invisibile che colpisce in maniera indiscriminata. di una guerra senza macerie visibili, ma con ferite profondissime che possiamo sanare solo con il tempo e il supporto di tutti. Non ci sono quindi le ragioni per contrastare questo scostamento che, come i precedenti, è stato concepito per sostenere la nostra sanità, le nostre famiglie, le nostre scuole e le nostre imprese. Gli italiani sono ottimisti di natura e noi abbiamo il dovere di agire per dare fiducia e sicurezza. Lo stiamo facendo e continueremo a farlo per il bene di tutti.

Signor Presidente, chiedo scusa per il ritardo, ma eravamo impegnati in una conferenza stampa con tutto il centrodestra. Ringrazio il Presidente, i colleghi che sono qui con noi e, soprattutto, il senso di responsabilità

sembra che alcuni dei punti sui quali Fratelli d'Italia e l'intero centrodestra si sono soffermati possano entrare a far parte della

L'attesa è verso l'interesse a superare la logica dei codici Ateco a favore di una logica della filiera, perché non ci sono figli e figliastri; ci sono lavoratori autonomi, imprese e partite IVA che hanno subito e subiscono cali di fatturato e fatturato e redditività e che devono tutti assieme essere considerati. Lo diciamo da mesi, pare che lo abbiate capito e ne siamo felici prima di tutto come italiani.

della destra, del centro e della sinistra del Parlamento italiano, dei rappresentanti dei cittadini. Pertanto, signor Presidente, avviandomi a concludere ritengo fondamentale garantire ai liberi professionisti italiani quell'attenzione che noi - lo ribadisco - abbiamo richiesto da mesi. Oggi mi rivolgo

adempimenti dichiarativi e questo rinvio delle scadenze fiscali. Ne abbiamo bisogno soprattutto noi italiani, ma ne hanno bisogno quei professionisti e quei commercialisti che stanno

risposta su questo e anche affinché ai professionisti vengano finalmente riconosciuti i ristori, perché sono esseri umani, lavoratori, sono il meccanismo principe della trasmissione delle regole dello Stato nell'economia. Aiutiamo anche loro come gli altri e quindi predisponiamo ammortizzatori sociali che valgano non solo per i lavoratori dipendenti, ma per tutti i lavoratori autonomi e i professionisti.

e si lasciò andare a tre affermazioni apparentemente granitiche: le scuole non chiuderanno, non verranno disposti nuovi *lockdown,* la condizione dell'economia italiana è quella di una vigorosa ripresa (uso le parole dello stesso Presidente del Consiglio). Chi aveva un minimo di conoscenza dei fatti e viveva nel mondo reale rimase sbalordito. Di lì a poco siamo precipitati nella condizione odierna: gli ospedali sono prossimi al collasso, abbiamo il *record* di morti per Covid-19, le previsioni di crescita sono ulteriormente calate, l'indebitamento è ulteriormente cresciuto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è nella condizione del mistero avvolto da un enigma e nessuno ne sa nulla. È evidente che questo Governo è inadeguato a fronteggiare la situazione è altrettanto evidente che viviamo in un momento di vera e propria tragedia nazionale. In condizioni del genere chi si trova all'opposizione ha due possibilità: la prima, la più comoda, è sedersi sulle rive del fiume e attendere che la corrente trasporti il cadavere politico del Presidente del Consiglio, del Governo, della maggioranza che lo sostiene. Si tratta di una posizione scivolosa e spiacevole nella misura in cui sappiamo tutti che, assieme al cadavere politico del Presidente del Consiglio, passerebbe anche il cadavere sociale della Nazione. fare proposte concrete, individuare problemi concreti e possibili soluzioni a problemi concreti senza nulla chiedere in cambio. Credo infatti e spero sia evidente a tutti che la questione dell'inciucio è una vera e propria infamia che non esiste nella realtà Silvio Berlusconi e Forza Italia hanno individuato nella metà del Paese che più sta pagando le conseguenze di questa crisi l'obiettivo politico da indicare al Governo: i non garantiti, le partite IVA, i lavoratori autonomi, quelli che più di altri sono oggi alle prese con il blocco totale delle proprie attività economiche. Il Governo ha accettato questa impostazione; ha accettato di farsi carico, come indicato dal nostro partito, di questa grave emergenza nazionale e sociale. Le opposizioni si sono giustamente allineate su una posizione di responsabilità

bisognerà che il Governo faccia in modo di restituire al Parlamento la propria funzione costituzionale di tutti gli atti emanati in questa crisi Covid. atti legislativi di iniziativa parlamentare sono il 10 per cento; il resto sono atti governativi o amministrativi. In tutta la storia del Governo Conte II è stato approvato l'1,03 per cento degli emendamenti presentati dal Parlamento, dai singoli parlamentari e dai Gruppi parlamentari. Non si può andare avanti così e non si può accettare il fatto che scelte decisive per il futuro del Paese vengano assunte dai tecnici del Ministero dell'economia e dai tecnici della Commissione europea nell'ignoranza del Paese e del Parlamento. Se vogliamo pensare di poter tirar fuori il Paese dalle secche nelle quali è finito, bisogna che tutti si assumano le proprie responsabilità. Bisogna che il Parlamento torni a essere centrale, che il narcisismo del Presidente del Consiglio e di altri *leader* venga accantonato; bisogna che tutti i partiti pensino non al proprio futuro, ma al futuro delle prossime generazioni sulle spalle delle quali stiamo gravando debiti potenzialmente insostenibili. In tempi non più facili rispetto a quelli che ci è dato vivere, quando la Nazione si dimostrò compatta e quando il ceto politico si dimostrò molto concreto, l'allora Presidente della Repubblica, il presidente della ricostruzione Luigi Einaudi, scrisse: «Nella vita delle nazioni di solito l'errore di non saper cogliere l'attimo fuggente è irreparabile».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Governo per la sua presenza. Arriviamo oggi all'ennesimo scostamento che, se vogliamo,

adesso sono arrivati tutti i vari decreti ristori con poca consistenza, salvo poi accorgersi che qualche consistenza ci doveva essere. Siamo al ristori-*quater*:

non dovevamo arrivare il 26 novembre a fare uno scostamento in fretta e furia perché vi siete accorti che il 30 novembre ci sono scadenze fiscali importanti. Autonomi, commercianti e artigiani il 30 novembre hanno gli F24 in scadenza. acconti sulle tasse per il 2020, ma se pensi di non aver fatturato puoi pagare l'80 per cento e non ti sanzioniamo. Insomma, gli autonomi devono avere davvero la sfera di cristallo per non incorrere in sanzioni. Poi cos'altro? Non lo so perché mi sono persa anch'io. La confusione è estrema ed è tanto più vergognosa perché siamo a ridosso delle scadenze.

se il commercialista è in quarantena e con lui tutto il suo ufficio, il contribuente è tenuto a fare da sé. Il contribuente deve sapere lui cosa pagare non è giustificato neanche per causa di forza maggiore. È così che ha risposto infatti l'Agenzia delle entrate ai tributaristi: non esiste nessuna impossibilità oggettivamente provata che giustifichi l'inadempimento.

Per favore, fate cancellare o rettificare urgentemente questa ignobile risposta che l'Agenzia delle entrate ha dato ai tributaristi.

e penso sia abbastanza vero. Abbiamo visto come ha affrontato l'epidemia, la pandemia, con i famosi DPCM, mai sufficienti e sempre intempestivi. Dal punto di vista economico, il Governo ha cercato poi di ridurre i danni e gli effetti economici negativi della pandemia, con i primi decreti-legge e poi con i ristori,

Sembra quasi che manchi quella famosa visione di cui parlavo in precedenza e l'impatto sociale è drammaticamente negativo, perché i garantiti sono già garantiti, mentre non lo sono coloro che garantiti non sono mai stati: mi riferisco agli autonomi, agli imprenditori, ai commercianti, ai precari, alle partite IVA, agli stagionali, ai consulenti, agli addetti del mondo dello spettacolo. La domanda, a questo punto, è se abbiamo la possibilità di avere veramente una visione rispetto a quanto ci è capitato. Probabilmente questa mancanza di visione si scontra con le nostre incapacità strutturali, con una inadeguatezza della classe politica, fondamentalmente, e con quei famosi lacci e lacciuoli, che hanno sempre bloccato anche i provvedimenti intempestivi che citavo in Forse manca anche una visione sui fondamentali di quello che accadrà dopo, alla fine di questa pandemia. Prima o dopo essa finirà, ma a quel punto ci sarà mancata quella visione, che dobbiamo anche proporre all'Europa e in base alla quale potremo trasformare e rivoluzionare il nostro Paese, come nel famoso dopoguerra. La capacità di visione appartiene tendenzialmente a quella categoria della politica che semplifica i problemi complessi. Si cerca di utilizzare una grammatica delle soluzioni immediate, senza infilarsi nei labirinti delle legislazioni successive e di quelle famose *matrioske*,

A mio avviso sarebbe stato molto meglio che tutte le risorse reperite a debito fossero state dedicate immediatamente a tutti coloro che hanno avuto una sofferenza economica a causa della pandemia. Faccio solo un esempio di carattere numerico:

Facciamo pure una tara del 30 per cento, rispetto ai 300 miliardi di euro, e arriviamo a 200 miliardi di euro, che sono più o meno la cifra degli scostamenti che sono stati deliberati. Sarebbe stato meglio? A mio avviso sì. seconda fase riguarda l'uscita dall'emergenza sanitaria. Abbiamo tamponato con difficoltà la prima e la seconda ondata, ma adesso ci aspetta uno straordinario piano vaccinale,

e con una seconda dopo diciotto giorni, ma anche con una anamnesi complessiva dei cittadini italiani, perché non si può inoculare loro il vaccino senza conoscerne lo stato clinico. Uno straordinario piano vaccinale che deve poi declinarsi nell'arco di due mesi, da metà gennaio a fine marzo, perché solo così si potrà raggiungere quella famosa immunità di gregge, o meglio di comunità, che potrebbe consentire oltre quel 15 per cento di italiani che hanno già contratto il virus. A questo siamo pronti? Siamo capaci? Ci sono anche le risorse finanziarie, il famoso MES: non volete prendere 37 miliardi, prendetene 20, ma con quei 20 mettete in piedi

a Bruxelles ogni tanto esagerano nel definire le pagelline e i tassi di democrazia interna di alcuni Paesi, anche perché quando Orban e Mateusz Morawiecki vanno ai Consigli di Stato e di Governo nessuno chiede loro la patente di democrazia: la tirano fuori solo quando c'è da dare i soldi, e guarda caso la Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe spesso sovrasta la legislazione nazionale. Non so se un Governo *pro tempore* riuscirà mai ad affrontare l'immane compito che lo attende. Penso che ci sia un'intera classe politica che si debba assumere questa responsabilità per dare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani nel 2030 un'Italia completamente diversa e rivoluzionata.

la pandemia in atto e le relative misure di prevenzione e contenimento stanno inevitabilmente innescando una crisi economica senza precedenti. In questo scenario, che vede coinvolti ampi settori produttivi e mette in sofferenza molte famiglie italiane, il voto favorevole all'ulteriore scostamento di bilancio richiesto oggi dal Governo risulta un atto dovuto, tant'è che prendo atto che nessuna delle opposizioni È chiaro, infatti, che in questo momento occorre prestare immediato soccorso a imprese, commercianti e lavoratori autonomi per evitare l'ulteriore impoverimento del tessuto produttivo nazionale e offrire aiuto concreto ai cittadini. Questo significa erogare indennizzi per chi ha dovuto chiudere la propria attività; significa integrare il fatturato di chi, pur non chiudendo, ha registrato sensibili contrazioni del proprio lavoro, posticipare le scadenze fiscali, erogare i sussidi di emergenza a chi non ce la fa. E tutto ciò va fatto subito. La strada imboccata dal Governo va ulteriormente percorsa con coraggio e determinazione, facendo ricorso a tutto il maggior indebitamento che sarà necessario. Questo, però, non vuol dire non scegliere con attenzione gli interventi da finanziare. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che i debiti che contraiamo oggi prima o poi dovranno essere ripagati e ricadranno sui nostri figli. Se è vero, infatti, che attualmente i nostri titoli di debito vengono acquistati dalla BCE, che potrà rifinanziarli e sterilizzarli per qualche tempo, tuttavia, non nutro alcuna fiducia sulla possibilità che tale debito pandemico venga annullato. Chi tira le fila della finanza europea e ha dettato i trattati ha scolpito nella pietra lo scopo ultimo del sistema bancario europeo, che è quello della stabilità dei prezzi, funzionale a non consentire la svalutazione dei crediti. Chi detiene le chiavi del sistema ha certamente interesse a finanziare gli Stati in periodi eccezionali come questi affinché il sistema europeo non si disgreghi, e tuttavia pretenderà sempre rigidi piani di rientro e non ha alcuna convenienza a rimettere i debiti ai propri debitori. Se è altresì vero che dall'anno prossimo potremo contare sui miliardi del *recovery fund*, è altrettanto vero che anche quelli sono, in definitiva, debiti dello Stato o dell'Unione europea che andranno ripagati o direttamente o indirettamente, attraverso la contribuzione al bilancio UE. In altre parole, non esiste alcuna pietra filosofale che crea l'oro dal nulla e non c'è a Bruxelles alcun benefattore che ci regala alcunché. Ogni centesimo che utilizzeremo oggi saremo chiamati a restituirlo domani come Nazione, con il sudore della fronte del nostro popolo. Questo introduce un tema di cui fino ad oggi non ho sentito discutere. Chi pagherà i costi di questa crisi? A chi intendiamo far ripagare, domani, l'ingente debito che siamo costretti a contrarre oggi? Già dalla legge di bilancio e dal piano nazionale, che dovrà decidere quali progetti finanziari realizzare con i 209 miliardi del *recovery fund*, occorrerà fare scelte politiche chiare, che non potranno accontentare tutti. Appena finirà lo stato di emergenza, occorrerà sostanziare il piano di rientro e mettere mano alla riforma fiscale operando scelte nette, che individuino chi e come dovrà pagare quanto spendiamo oggi. La crisi e la necessità di reperire le risorse per pagare i debiti e di selezionare i progetti su cui investire rendono, a mio giudizio, non percorribile il percorso di larghe intese di cui sento parlare e vagheggiare molti. Su questi temi, il MoVimento non può trovare punti d'intesa con Forza Italia: riteniamo che sia somma ingiustizia trattare ugualmente situazioni diseguali, pertanto proponiamo la progressività della tassazione, per far pagare di più chi ha di più; Forza Italia, al contrario, vorrebbe moratorie generalizzate, in cui i soliti furbi possano confondersi con i bisognosi, e far pagare poco anche a chi ha tanto, con la conseguenza inevitabile di far pagare di più a chi ha meno, oppure di tagliare i servizi pubblici. Il nostro MoVimento è nato affinché ciascun cittadino contasse come gli altri; il vostro partito affinché le *élite* contino di più delle masse. Noi vogliamo che le leggi siano uguali per tutti e aspiriamo a fare leggi utili ai più; Forza Italia non si fa scrupoli a fare leggi *ad personam*, com'è già avvenuto in passato, finalizzate all'interesse di pochi a scapito di molti. Noi vogliamo combattere con rigore l'evasione fiscale, mentre Forza Italia ha il proprio *leader* condannato per frode fiscale. Noi vogliamo la legalità e vogliamo sradicare la criminalità organizzata e l'economia ad essa collegata, che soffoca le imprese sane, mentre Forza Italia

sarebbe utopico, errato e foriero di gravi equivoci scrivere assieme la legge finanziaria, il piano nazionale di ripresa o la riforma fiscale. Vi voglio fare un esempio concreto. Due economisti francesi, nel libro «Il trionfo dell'ingiustizia», dimostrano che oggi nel mondo le diseguaglianze sono aumentate e che proprio nei periodi di periodi la ricchezza tenda ad aumentare in poche mani; aumenta la povertà di molti, ma anche la ricchezza di pochi. Questo libro dimostra anche che i ricchi pagano meno tasse dei poveri e come sia invece doveroso e possibile costruire un sistema fiscale che riduca le disuguaglianze e, in definitiva, costruisca un mondo più equo. Seguendo tali teorie, se si applicasse un prelievo del 2 per cento ai circa 3.000 italiani che hanno oggi una ricchezza superiore ai 50 milioni di euro per cento ai circa 40 soggetti con ricchezza superiore al miliardo di euro, si ricaverebbe un contributo di emergenza di circa 10 miliardi, che potrebbe essere utilizzato a beneficio dei bisognosi e delle classi medie, sempre più provate dalla crisi. Queste proposte, così come quella della minor tassazione dei redditi da lavoro rispetto alle rendite da capitale, potrebbero certamente essere portate avanti dal MoVimento 5 Stelle, ma credete che possano essere condivise da forze conservatrici come Forza Italia? Per questi motivi, voterò a favore dello scostamento di bilancio richiesto dal Governo, ma ammonisco al contempo i colleghi di maggioranza a non intraprendere strade che ci svierebbero dagli obiettivi di cambiamento e di equità che il Paese necessita e pretende.

mi ha stimolato innanzi tutto un quesito: che senso ha fare politica? Qual è la ragione per cui siamo qui a rappresentare il popolo? Per erigere muri e catturare qualche *like* oppure per cercare di portare il nostro contributo, che si fonda sulla nostra storia, sulla nostra cultura e sui nostri valori? signor Presidente, lei è una persona sensibile anche alla storia del nostro Paese. Si immagini se dopo le macerie della seconda guerra mondiale questo Parlamento avesse posto in essere una tale dialettica, perché di questo stiamo parlando. Noi siamo quelli che alla Conferenza di Parigi hanno fatto leva solo sulla cortesia personale degli altri *leader* dei Paesi stranieri

politici: e tutto questo è stato possibile perché c'erano uomini e donne che hanno avuto lungimiranza e hanno costruito ponti, non che hanno denigrato l'avversario solo ed esclusivamente per un tornaconto personale. Noi siamo questo. *(Applausi)*. Siamo quelli che hanno difeso la democrazia e permettiamo a un senatore del del Parlamento di dire cose del tutto infondate. Siamo quelli che hanno difeso la proprietà privata e la libertà in questo Paese, quindi non prendiamo lezioni da chi oggi ha il solo scopo di dividerlo durante una delle sue più grandi tragedie dalla nascita della Repubblica. Non credo,

Bisogna esserlo, però, uomini di Stato, che mettono al servizio del Paese la propria cultura, i propri valori e la propria formazione. E allora lo dico, signor Presidente: oggi non vince una parte politica al Governo e neanche l'opposizione; oggi vince il Paese, e lo dobbiamo dire con l'orgoglio di questo Parlamento troppe volte denigrato all'esterno di questo palazzo. Oggi vince il Paese, perché credo che anche noi, come opposizione, stiamo cambiando paradigma:

non ho nulla da dire né da insegnare a nessuno. Dico solo che in politica mi hanno insegnato una regola: il rispetto degli altri e delle idee diverse dalle mie, quindi non cado nella trappola di chi oggi pensa solo a offendere. *(Applausi)*. Signor Presidente, potendo concedermi il lusso di sottrarmi da questa discussione un po' imbarazzante, tale per cui, mentre votate insieme, vi insultate, vorrei tentare di riportarla di riportarla sul terreno del merito, perché +Europa-Azione ha votato convintamente i primi scostamenti di bilancio. Lo abbiamo fatto nella consapevolezza e nella convinzione che far fronte all'emergenza, sia sanitaria sia economica, fosse una responsabilità che non attiene alla sola maggioranza e al solo Governo, per cui abbiamo accolto i primi inviti del Governo Conte a votare in maniera condivisa. Insieme a quella disponibilità al voto, abbiamo offerto al Governo anche qualcos'altro: proposte puntuali e collaborazione su questioni specifiche. Ne ricordo solo alcune, perché purtroppo sono ancora di drammatica attualità. Avevamo proposto al ministro Gualtieri la restituzione dei versamenti degli acconti IRES e IRAP, per dare immediato e proporzionato ristoro alle imprese, oltre che un intervento molto veloce nelle casse delle aziende. Avevamo proposto al ministro Speranza e al ministro Manfredi il finanziamento di tutte le borse di specializzazione in medicina, per superare l'ormai annoso problema dell'imbuto formativo. celebriamo le nuove larghe intese, fuori ci sono ragazzi che da mesi - da settembre ormai, e siamo a dicembre - aspettano di sapere il loro destino circa l'esame per l'accesso alla specializzazione. Lo dico fuori da ogni polemica, perché si parla di emergenza, di sanità e di medici e faremmo bene a tenerne conto. Abbiamo chiesto al ministro Speranza, con una risoluzione che è stata bocciata, è stata bocciata, un rendiconto puntuale dei 9 miliardi fin qui destinati alla sanità, senza nessuna polemica, perché, se ci si chiede di condividere una decisione, condividiamo anche se l'utilizzo delle risorse è funzionale ed efficiente o meno. Abbiamo proposto al Governo a maggio, molto prima dell'estate, il cosiddetto piano a semafori, una riapertura graduale grazie alla quale, che se forse l'avessimo utilizzata quest'estate, non saremmo nelle condizioni attuali. attuali. A più riprese, su iniziativa della senatrice Bonino, abbiamo chiesto a quest'Assemblea di esprimersi, non per un capriccio né per uno sfizio europeista, sulla questione del MES disponibile da giugno, perché sta diventando insopportabile ogni giorno leggere la cronaca che racconta di tamponi insufficienti, corsa agli ospedali da campo, personale sottoposto a turni esasperanti e prestazioni in difficoltà. Se non si è d'accordo, lo si dica: da mesi state sottoponendo questo Parlamento, dentro le tecnicalità regolamentari, di fronte all'impossibilità di esprimersi sul punto. Poiché la gravità della situazione impedisce a ciascuno di noi, me compreso, il ricorso alla polemica e all'atteggiamento di non disponibilità, vorrei chiedere al Governo, signor Presidente, su cosa ci viene chiesta collaborazione. Su cosa dovremmo condividere l'azione di Governo? Sulle nomine del commissario alla sanità in Calabria? Con quale Governo dovremmo collaborare? Con quello che questa mattina, per voce del ministro Speranza, ha detto che il MES è indispensabile o con quello che, per voce del ministro Di Maio - entrambi rispettabili - dice che non se ne parla proprio? Prima di fare appelli alla collaborazione e all'unità, dovreste fare chiarezza, perché questa sera,

scorre sotto, chiedendo ai medici di rendersi disponibili perché c'è un'emergenza in atto e non ci sono abbastanza medici, e noi continuiamo a dire di no a risorse destinate alla sanità. Per tali ragioni, invitateci quando volete sollevare il Paese, non quando volete metterlo definitivamente in ginocchio. la relazione in esame accompagna il quinto scostamento di bilancio, un'operazione tutta costruita sul 2020, inedita per il nostro Paese: non c'è memoria nell'articolazione della Repubblica della gestione di una fase così complessa

Voglio dire immediatamente che ci sentiamo responsabili e condividiamo l'impianto valoriale che il Governo ha assunto per affrontare l'emergenza, nei suoi princìpi fondamentali: proteggere il lavoro; non lasciare nessuno nella solitudine; favorire la liquidità delle imprese, che sono un patrimonio del nostro Paese e della nostra comunità

Lo dico ai colleghi dell'opposizione: dobbiamo renderci conto, prima di tutto tra di noi, di essere all'interno di una fase emergenziale che attraversa l'Europa il mondo nella sua interezza e cambierà di molto le dinamiche economiche e sociali delle nostre comunità. comunità. Ci sentiamo rappresentati dalle misure che il Governo ha introdotto per attraversare questa crisi, perché dobbiamo fare un salto di qualità nel tenere insieme la gestione dell'emergenza con un più preciso progetto per uscire dall'emergenza stessa e dalla crisi. Abbiamo bisogno, cioè, di affiancare a questi principi e a questi valori condivisi un'idea più precisa di come usciremo dalla crisi e sarà un'uscita diversa. motivo che trovo che i luoghi comuni al passato non siano più nelle condizioni di rappresentare il futuro. *(Applausi)*. Per abitare il futuro non serve

il mercato e lo Stato. Questa crisi ci mostra un'esigenza nuova: il lavoro e il capitale sono più vicini e non più lontani del passato hanno bisogno di iniziative riformiste nuove per poter unire e non dividere; abbiamo bisogno di superare le dietrologie del passato, perché per noi le partite IVA e il lavoro autonomo non sono un retaggio di elusione ed evasione fiscale, ma un pezzo fondamentale dell'intraprendere, necessario per portare il Paese fuori dalla crisi, per costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. - e mi rivolgo innanzitutto al Ministro e alla maggioranza - che abbiamo bisogno di precisare meglio il nostro profilo di Paese in uscita dalla pandemia. Questo non significa che non ci sia spazio per migliorare in termini di efficienza ed efficacia: i decreti ristori nascono per dare una risposta immediata e tempestiva a dinamiche economiche che peraltro, rispetto alla prima ondata, nella seconda sono ancora più complicate, perché

che intraprendere la professione sanitaria e medica non è una scelta che spinge alla solitudine, ma risponde alla straordinaria necessità di portare nella medicina territoriale, cioè a casa delle persone, il diritto alla salute. Non possiamo affermare un giorno che per uscire dalla crisi la prima risposta dev'essere di carattere sanitario, cioè mettere in sicurezza il diritto alla salute, e non avere un progetto più preciso e più puntuale su come ristrutturare il sistema sanitario. Questo è il motivo per il quale possiamo attrarre le risorse europee. Se abbiamo un progetto, dobbiamo attrarre le risorse europee. Non dobbiamo avere difficoltà a discutere in termini ideologici sul nuovo volto dell'Europa, ma prima dobbiamo indicare con chiarezza dove servono le risorse, dove vanno utilizzate e cosa migliora in termini di diritto alla salute per i nostri cittadini. Questo è il primo passaggio da compiere. Il secondo è che dobbiamo approfittare di quel nuovo volto dell'Europa. Ricordo che questa legislatura, purtroppo, iniziò sul no all'Europa, no all'euro, sul no alla scienza e, in molti casi, anche con una contrapposizione sui temi delle vaccinazioni. Penso che oggi ci rendiamo conto tutti di quanto servano non solo l'Europa, anche la scienza e la conoscenza. Grazie alla scienza, infatti, riusciremo a garantire a tutti i cittadini italiani un'uscita dalla pandemia. Abbiamo capovolto tutto questo. Ne siamo orgogliosi. Ecco perché penso che occorra accelerare sull'idea di come usare da questa crisi e di quale profilo economico e sociale offrire agli italiani per dare una risposta di sicurezza, in quanto recuperare i termini della fiducia è indispensabile per le nuove dinamiche economiche. Abbiamo bisogno di accelerare gli investimenti. Non compiamo errori, pensando di fermarci ai progetti. Dobbiamo entrare nel merito del processo per realizzare un investimento. Si devono ridurre i tempi. Ecco che le nuove dinamiche europee devono anche offrirci le condizioni per ritornare a dare valore alla pubblica amministrazione, alla pubblica amministrazione, che deve migliorare in efficienza e in competitività, ma deve tornare a essere una bella parola, non un centro di spreco e di costo: è la più grande e più importante necessità che abbiamo per dare velocità ai processi ed efficienza alle procedure. C'è differenza: come un vaccino non è la vaccinazione, così un progetto non è l'opera pubblica realizzata; lì in mezzo c'è il ruolo dello Stato, che dev'essere nelle condizioni di garantire efficacia ed efficienza. Prendo atto con grande favore dell'indirizzo che ho visto: il passaggio, cioè, dal voto di astensione di ieri in Commissione da parte del centro destra a quello favorevole di oggi alla Camera. È il segnale che le nostre idee, che richiamavano ad unità e responsabilità nell'interesse generale del Paese, hanno trovato finalmente un percorso corretto. È un bel passaggio, quello dall'astensione di ieri in Commissione al voto favorevole di oggi: significa che questa volta vincono l'Italia e la responsabilità nazionale.

dopo l'ultimo scostamento di circa 22 miliardi di euro, oggi non ci fosse più bisogno di questo strumento di indebitamento, anche perché il Governo, in quell'occasione, ancora una volta ci aveva assicurato

per sostenere, in questo momento particolare, i redditi dei commercianti, degli artigiani, delle aziende, dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura del nostro Paese. miliardi di euro per provvedere a un nuovo decreto ristori; abbiamo fatto il primo, il secondo, il terzo e il quarto: noi, ancora una volta, non condividiamo questo modo di fare provvedimenti "a spezzatino"; quello che abbiamo sempre chiesto e che abbiamo offerto come collaborazione al Governo è di avere invece una visione

Ci siamo imposti, come forze politiche di centrodestra, per chiedere appunto

in questi mesi ha distrutto il tessuto produttivo del nostro Paese, che - come dicevo - si regge sulle piccole e medie imprese, sull'artigianato, sul commercio e sui liberi professionisti. A loro e solo a loro devono essere destinate oggi queste risorse; a queste categorie

è stata perseguita. Non ci fermeremo qui. Adesso si apre il dibattito sulla manovra finanziaria, che è importante proprio per guardare alle nuove generazioni e al futuro del nostro Paese. Continueremo a perseguire la via migliore, nel solo e unico interesse del Paese. Signor Presidente, il Governo ci chiede ancora una volta di esaminare la richiesta di uno scostamento di bilancio, oggi di 8 miliardi.

la domanda a cui credo che tutti dobbiamo rispondere è principalmente questa: lo scostamento è necessario? È utile al Paese? È determinante per dare risposte alla grave crisi che stiamo affrontando? Tali domande hanno una sola risposta ed è affermativa: lo scostamento è assolutamente necessario. Il tema di fondo però, abbiamo sempre sottolineato, non è tanto fare indebitamento. È ovvio che è un danno per i bilanci e per il futuro del nostro Paese indebitarsi per queste somme così ingenti, ma è il periodo drammatico che stiamo vivendo a richiederlo. Noi però abbiamo sempre posto un tema: come si spendono questi soldi? *(Applausi)*. L'abbiamo posto sin dalla prima volta e abbiamo da subito cercato di dare il nostro contributo, ma, al di là di una disponibilità di facciata, sia nelle Commissioni, sia a livello di Governo, la risposta è sempre stata elusiva; non abbiamo mai avuto la soddisfazione di vedere accolte le nostre proposte e neanche di vederle prese in considerazione. La sensazione è che avete sempre fatto finta di volerci ascoltare e di aprire un dialogo, esclusivamente per dare al Paese una bella sensazione e una bella immagine del vostro atteggiamento che era fatto però di finzione e falsità, che purtroppo appartiene a molti esponenti del vostro Governo, *in primis* - permettetemelo, questa è la mia sensazione e la mia convinzione - al vostro Presidente del Consiglio. bella immagine di facciata, ma nella sostanza non ci sono nulla di buono per il Paese né nulla di utile al confronto con le opposizioni. È necessario, questo scostamento, perché nel giro di poco meno di trenta giorni avete approvato quattro decreti ristoro, a dimostrazione della vostra approssimazione, della mancanza di strategia, della mancata comprensione della gravità della situazione che stiamo vivendo, in un'eterna rincorsa ad affrontare i problemi economici del Paese. Questo stato confusionale del Governo non ce lo possiamo permettere e non potevamo permettervi di procedere a un piano ristori basato sui colori delle Regioni: è inaccettabile. No ai ristori in base alle zone rosse, arancioni e gialle, che variano di settimana in settimana. No alla lotteria dei colori; sì invece in base al calo del fatturato: questo è il criterio di base giusto e sacrosanto che dev'essere utilizzato da Nord a Sud Regioni gialle, rosse, arancioni e di tutti i colori che volete attribuire agli enti territoriali. È l'unico criterio che può essere utilizzato e sul quale anche anche in Commissione abbiamo insistito. Questo sarà il banco di prova: se utilizzerete questo criterio, evidentemente non potrete che avere la nostra approvazione nei prossimi provvedimenti. Se così non fosse e per l'ennesima volta ci prenderete in giro, credo che questa sarà l'ultima in cui potremo partecipare all'assunzione di responsabilità di procedere agli scostamenti di bilancio. Questo scostamento è assolutamente necessario, perché negli ultimi mesi vi siete dimenticati totalmente del dramma che stanno vivendo lavoratori autonomi, partite IVA, artigiani, commercianti, imprenditori e lavoratori stagionali senza occupazione. Tutti stanno subendo i danni di questa pandemia da un punto di vista sanitario, emotivo e psicologico, ogni cittadino di questo Paese e ogni cittadino del mondo; a livello economico è innegabile però che qualcuno li stia pagando più di altri. Non ho mai creduto e - neppure - la Lega alle contrapposizioni tra dipendenti pubblici, lavoratori autonomi e dipendenti privati: siamo tutti sulla stessa barca, soprattutto in un momento così drammatico, dobbiamo un grazie a tutti i dipendenti pubblici che stanno garantendo i servizi fondamentali al nostro Paese, dalla scuola alle Forze dell'ordine in particolare e alla sanità pubblica, che sono sotto pressione giorno per giorno e sul fronte. *(Applausi)*. A loro va il nostro grazie incondizionato, ma è innegabile che da un punto di vista economico qualcuno abbia lo stipendio garantito (almeno quella sicurezza ce l'ha) e qualcun altro invece sia in crisi nera e totale ormai da mesi mesi e non possa più reggere a quello che stiamo vivendo. *(Applausi)*. È per questo che abbiamo insistito sin dall'inizio che gli interventi fossero indirizzati a queste categorie, a chi produce ricchezza e lavoro, paga le tasse (sproporzionate, ma le paga) e cerca di onorare il proprio ruolo di contribuente, ma in questo momento è ormai al limite. Vi chiediamo anche un intervento a livello europeo per garantire equità nella gestione della stagione turistica invernale. Guardate che sulle nostre montagne o si permette di lavorare o, anche lì, dovranno essere garantiti indennizzi per tutti. Il tema di fondo - e qui l'ironia proprio non serve - non è se fare le vacanze o andare a sciare; il tema sono le aziende che

di fronte a questa necessità dovete dare una risposta e dovete farlo a livello europeo. Il Paese sta soffrendo e voi agite sempre in ritardo, in affanno e senza una strategia chiara.

- permettetemi - è ancora più drammatico che il Governo l'abbia nominato e che, a distanza di giorni, non abbia ancora trovato un sostituto degno di questo nome. *(Applausi)*. Siete complici di quel commissario e dei suoi ritardi

Noi faremo la nostra parte, come abbiamo sempre fatto. Questo non è il primo scostamento di bilancio che ci troviamo ad affrontare; sapete che li abbiamo sempre approvati, garantendo il nostro voto, che, in un caso, è stato anche determinante. Infatti, necessari, almeno in un'occasione, sono stati garantiti dal centrodestra e dal nostro senso di responsabilità nei confronti del Paese. Non abbiamo mai ostacolato l'attività di Commissione e Assemblea e abbiamo dato il nostro contributo.

e necessario per superare questa crisi senza precedenti. La Lega c'è e farà la propria parte, insieme al centrodestra; non ci sottrarremo mai al confronto e ci assumeremo sempre le nostre responsabilità. In conclusione, cambiato atteggiamento, come ha voluto dire il collega Manca. Il nostro atteggiamento non è mai cambiato ed è sempre stato coerente: avanzare proposte,

sconfinata di partite IVA, autonomi, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori e tutti i lavoratori dipendenti e stagionali che lavorano per loro sia garantita da un Esecutivo che fino adesso, per loro, ha fatto poco o niente. *(Applausi)*.

alla questione dei ristori e dei tanti sostegni che il Governo ha messo coraggiosamente in campo in questi mesi, anche per quanto riguarda il settore dello spettacolo dal vivo, per esempio, è emersa la problematica legata ai codici Ateco. Anche da Anche da lì è arrivata la richiesta di valutare il passaggio a un'ottica di filiera. Infatti, se i codici Ateco potevano essere utili nel quadro emergenziale e nella necessità di provvedere a sostegni economici nei tempi

sostegni arrivino effettivamente a tutta la platea di lavoratori e imprese - che esistono anche nel mondo dello spettacolo e della cultura - che necessitano di un sostegno. assolutamente di non dimenticarci dei teatri privati, che svolgono una funzione assolutamente essenziale, non solo per dilettarci nel tempo libero, ma anche per tutto quello che il teatro ci insegna ogni volta che ci mettiamo piede, in termini di lettura di noi stessi, della società e del tempo in cui viviamo. Accanto a questo, vorrei richiamare l'attenzione anche su alcune richieste più strutturali che sono arrivate, ovvero l'estensione dell'art bonus e dei crediti d'imposta e la defiscalizzazione dei consumi culturali, proprio perché consumare cultura consumare cultura è un bene essenziale e, come tale, va trattato e dobbiamo favorirne la fruizione il più possibile, soprattutto tra le fasce meno agiate. dunque, infine, anche a una rimodulazione di alcune aliquote IVA e a un'estensione di alcuni crediti di imposta, perché ci sono settori che ancora non godono di questa misura. vorrei passare anche a quella che io reputo essere la situazione più cogente: quella cioè che riguarda lo spettacolo dal vivo e i suoi lavoratori, perché, come non mi stancherò di ripetere, in questa fase pandemica è emersa la drammaticità dell'inesistenza di un sistema di *welfare* dedicato *ad hoc* a questi lavoratori che non hanno

Gribaudo e Carbonaro che hanno depositato un disegno di legge. A questo proposito apro una parentesi: dobbiamo assolutamente continuare a portare avanti i lavori parlamentari nelle Commissioni,

ed è questo il momento perché il tempo stringe. La Costituzione prevede infatti che una legislatura duri cinque anni (non lo abbiamo deciso noi in questa maggioranza), dunque tutti noi avremmo piacere di arrivare a scadenza della legislatura

hoc* per i lavoratori dello spettacolo, ma occorre anche riprendere l'esame del disegno di legge collegato sullo spettacolo dal vivo

rispetto alle risorse che decidiamo di impiegare nella legge di bilancio, all'ambiente e alla cultura ancora spetta una fetta da pulcino. Non dovrebbe essere così, perché oltre alla crisi sociale che seguirà questa crisi pandemica ci sarà anche la crisi climatica la crisi climatica che è destinata ad impattare anche sui nostri beni culturali. Io sono qui oggi perché i lavoratori dello spettacolo devono essere rappresentati in questa sede e noi dobbiamo essere la loro voce; dobbiamo però essere ancora di più la voce di chi non ha voce, cioè di tutto il nostro patrimonio artistico e architettonico che non ha voce, ma che ci narra la nostra storia,

diede una martellata a una sua scultura chiedendole di parlare; allora io oggi mi prendo l'onere di parlare per quel patrimonio e di chiedervi di non dimenticarlo. Qualche giorno fa, a proposito dell'anniversario del sisma dell'Irpinia, è stata riproposta un'intervista che Lina Wertmüller fece a Martin Scorsese,

non torneranno più in quei luoghi, sapere che quei luoghi mantengono intatta la loro bellezza, sapere che c'è ancora quel monumento, che c'è ancora quella bottega - mi riferisco all'artigianato e ai nostri saperi - che ci sono ancora quel cinema e quel teatro

Presidente, dal dibattito emerge un indirizzo importante che viene dato al Governo per poter procedere con questo nuovo scostamento, con finalità che sono state chiarite dai diversi Gruppi e che mi auguro il Governo possa prendere in considerazione in maniera ampia ed esaustiva, proprio per dare soddisfazione al Parlamento stesso. Se è possibile avere i testi delle proposte di risoluzione presentate, possiamo anche esprimere il parere.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Signor Presidente, ringrazio le senatrici e i senatori intervenuti nel dibattito su un passaggio particolarmente significativo delle scelte di politica economica e finanziaria. Non a caso, l'articolo 81 della Costituzione prescrive per le votazioni sugli scostamenti di bilancio non l'approvazione a maggioranza semplice, ma a maggioranza dei componenti della Camera e del Senato della Repubblica. La *ratio* di questo dell'articolo 81 è, di fatto, un invito alla ricerca di un'ampia condivisione in Parlamento su scelte che implicano conseguenze che impattano non solo sul presente, ma anche sulle generazioni future. infatti, di richieste di indebitamento che si traducono in maggiore debito pubblico. La richiesta di maggiore indebitamento segue le analoghe richieste votate dal Parlamento da marzo in avanti, come veniva ricordato. La prima era di 20 miliardi di euro, la seconda di 55 miliardi di euro, la terza di 25 e quest'ultima è di 8 miliardi e porta il totale di autorizzazioni richieste dal Governo al Parlamento a 108 miliardi di euro. È un ammontare senza precedenti; è l'equivalente di cinque leggi di bilancio, come è stato ricordato anche nel dibattito odierno. È un ammontare di risorse straordinariamente elevato di fronte a una situazione eccezionale dal punto di vista sanitario, economico e sociale. La pandemia ha investito per prima l'Italia in Europa con una prima ondata terribile nei mesi di marzo, aprile e maggio. Da qualche settimana l'Europa e anche il nostro Paese devono fronteggiare una seconda ondata, che stiamo affrontando con misure restrittive dolorose, diverse da quelle che fummo costretti ad adottare ad inizio marzo. Infatti, nel frattempo abbiamo costruito e condiviso con le Regioni un sistema di monitoraggio, che non avevamo a disposizione all'inizio della pandemia e che oggi ci ha permesso di differenziare dal punto di vista territoriale, in relazione alla gravità, Regione per Regione, dei dati epidemiologici e ci ha permesso di limitare, parzialmente o totalmente, l'attività di alcuni settori economici, mantenendo aperta la gran parte delle attività economiche del Paese, a differenza delle misure fortemente restrittive, che fummo costretti ad adottare Questo nuovo modello di misure di sicurezza, che abbiamo adottato a partire dai DPCM di fine ottobre e soprattutto di inizio novembre, sta producendo alcuni primi risultati positivi. sottolineare che va mantenuto un principio di massima cautela e di prudenza, ma i dati, che quotidianamente vengono forniti e valutati dalla cabina di regia, indicano che non c'è più la crescita esponenziale dei contagi e della pressione sul sistema ospedaliero, che registravamo fino a pochi giorni fa. che dobbiamo fare i conti con le conseguenze economiche delle misure restrittive, che sono state adottate per fronteggiare questa seconda ondata. Sono conseguenze economiche, come ha indicato il Ministro dell'economia e delle finanze, ma anche la Banca d'Italia nella sua audizione, meno pesanti rispetto a quelle che l'economia ha sofferto da marzo in avanti, ma sono comunque conseguenze economiche significative e particolarmente dolorose per le attività economiche direttamente coinvolte dalle misure restrittive. È a questo scopo che abbiamo via via adottato tre decreti ristori, che sono all'esame del Senato della Repubblica. Abbiamo adottato una sequenza di provvedimenti, perché abbiamo cercato di costruire un meccanismo di sostegno e di ristoro, che tenesse conto di questo nuovo modello di contenimento della pandemia, differenziato per settore economico e per territorio. Questi tre decreti hanno messo in campo risorse, che hanno superato largamente la cifra di 10 miliardi di euro. È evidente però che quelle risorse non sono sufficienti ad affrontare e a ristorare, per quanto necessario, le attività economiche interessate da queste misure restrittive ed è per questo motivo, per sostenere fino in fondo chi è impattato dalle misure restrittive, che il Governo oggi chiede un nuovo scostamento di 8 miliardi di euro. Ho registrato con grande apprezzamento il clima e i contenuti di condivisione venuti dalle forze di maggioranza e dalle forze di opposizione, nei confronti di questa richiesta del Governo. tratti di un passaggio molto importante dal punto di vista politico, che risponde positivamente ai richiami del Capo dello Stato e alle attese da parte del Paese di una risposta corale della politica, che non cancella le differenze di valutazione e di proposta delle forze di opposizione, nei confronti del lavoro che il Governo ha messo in campo in questi mesi, ma che

che c'è stata in questi giorni con le forze di opposizione per un utilizzo di questi 8 miliardi di euro; l'interlocuzione che raccoglie la sensibilità espressa da tutte le forze parlamentari, in particolare anche da quelle di opposizione, nei confronti di un intervento che risponda a quella parte del Paese che fa impresa, che svolge il proprio lavoro in modo autonomo e indipendente,

in questo Paese, ma altresì di lavorare con tutti gli strumenti di sostegno che possiamo mettere in campo per tenere assieme questo Paese, per tenerlo coeso in una fase particolarmente difficile. È per questo che dedicheremo la quasi totalità delle risorse a un intervento sul terreno fiscale, per rinviare le scadenze fiscali previste dal 30 novembre in avanti, il secondo acconto Irpef, Ires e Irap, i versamenti IVA, i versamenti dei contributi, i versamenti delle ritenute, naturalmente privilegiando chi subisce significativi cali di fatturato. Abbiamo infatti il dovere di essere selettivi e di utilizzare le risorse dei contribuenti - che in questo caso chiediamo al Parlamento - per aiutare chi è maggiormente in condizioni di bisogno. Costruiamo un intervento che guarda anzitutto a quella parte del Paese utilizzando lo strumento del rinvio di questi versamenti. che si è riflessa nei contenuti delle risoluzioni presentate al Parlamento, chiama in causa anche il meccanismo dei ristori. In questa fase abbiamo costruito ristori sulla base dei codici Ateco perché questo era lo strumento per fare arrivare il più rapidamente possibile le risorse alle attività direttamente impattate in assenza dei dati di fatturato. Oggi, infatti, non abbiamo i dati aggiornati che ci permettano di capire chi nel mese di novembre - quando sono partite le misure restrittive - ha avuto perdite di fatturato e chi no. no. È per questo che abbiamo costruito un meccanismo che partiva dal contributo a fondo perduto, definito con il decreto-legge rilancio, dando risorse ulteriori alle attività direttamente interessate. Un meccanismo sicuramente imperfetto, ma che è stato scelto per la rapidità Ieri l'Agenzia delle entrate ha comunicato di avere completato il versamento dei ristori a tutte le attività, a tutti i codici Ateco individuati dal primo decreto-legge ristori, e nei prossimi giorni questi contributi saranno seguiti dalle categorie, dalle attività individuate dai provvedimenti successivi. È evidente, però, che noi - ragionando in una prospettiva che non riguarda direttamente questo scostamento - dobbiamo immaginare per l'immediato futuro un meccanismo più generale di sostegno al mondo del lavoro autonomo, delle piccole e medie imprese, dei liberi professionisti, delle partite IVA; che guardi a quello che è accaduto effettivamente in questi mesi (e questo lo sapremo, però, non adesso, ma a partire da gennaio) e che preveda una forma di sostegno significativo nei confronti di questo pezzo cruciale del mondo del lavoro italiano che non può contare sulla cassa integrazione né su strumenti di protezione sociale che invece tutelano il lavoro dipendente, per come è organizzato oggi il nostro modello di *welfare*. Queste sono

di prospettiva su cui rinnoviamo l'invito al dialogo a tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, per proseguire - è l'auspicio che mi sento di fare in questa sede - un percorso di condivisione dello sforzo della politica economica di sostegno nei confronti delle imprese e delle famiglie che dovremo proseguire anche nei prossimi mesi. Colleghi, sono arrivate notizie positive sul fronte della ricerca sui vaccini, che vede l'Unione europea e l'Italia con un ruolo da protagoniste. Il ministro Speranza il 2 dicembre presenterà al Parlamento il piano di distribuzione dei vaccini nel nostro Paese, ma dovremo stringere i denti ancora per molti mesi. Abbiamo il dovere di fare un discorso di verità agli italiani e di assumerci la responsabilità, sul fronte della politica economica, di proseguire le misure di sostegno alle imprese e alle famiglie che guardano all'emergenza. Contemporaneamente - ma questo lo faremo innanzitutto nella discussione sulla legge di bilancio - dobbiamo costruire un progetto di medio-lungo periodo Questo è il lavoro che siamo tutti chiamati a fare in questa fase difficile della vita del Paese e sono molto contento che da tutti i Gruppi parlamentari anche in Senato sia venuta una risposta positiva

Presidente, credo che il vice ministro Misiani abbia fatto una descrizione molto precisa e puntuale del lavoro condotto in questi mesi e anche delle ragioni che hanno ispirato il Governo a richiedere questo nuovo

queste risorse prioritariamente a chi ancora non aveva avuto adeguati ristori, quindi il mondo delle partite IVA, dei lavoratori autonomi e dei commercianti. Il Governo mi sembra abbia recepito l'invito arrivato da tutte le forze politiche che siedono in Parlamento quindi, rispetto ai testi delle proposte di risoluzione che sono state presentate

Signor Presidente, colleghe e colleghi, come è stato sottolineato in Commissione, i dati negativi di queste settimane vengono compensati dal forte rimbalzo congiunturale dei mesi estivi. Ci si è domandati se fosse davvero necessario un ulteriore scostamento di 8 miliardi a fronte di un quadro sostanzialmente identico a quello previsto dalla Nota di La risposta è che la nuova ondata della pandemia inciderà negativamente sul 2021 con un rimbalzo del PIL che non supererà il 5 per cento. L'altro elemento si chiama quella sui tempi dell'erogazione delle risorse del *recovery fund* e quella sui tempi di contenimento della pandemia con l'arrivo del vaccino. Pertanto, questo scostamento risponde a un principio prudenziale che per noi è assolutamente condivisibile; non sarà per certo l'ultimo. Il comparto produttivo durante i mesi estivi ha mostrato una resilienza che ci deve incoraggiare per il futuro, a condizione che si compiano scelte adeguate. oggi il tema è quello del rapporto col fisco di cittadini, liberi professionisti e imprese. Dobbiamo mettere in campo strumenti per non mandare le imprese in crisi di liquidità, aiutandole anche a chiudere i vecchi contenziosi, con stralcio di interessi, moratorie e rinegoziazione dei debiti soprattutto per le piccole cartelle, sospensione dei pagamenti e proroga delle scadenze, a cominciare da quelle previste da qui alla fine dell'anno. Fatemi aprire una piccola parentesi. Le imprese, i commercianti, gli artigiani, i lavoratori autonomi e le partite IVA stanno soffrendo tremendamente anche per i divieti di attività imposti con i DPCM, imposti con i DPCM, pur giusti. È il momento di imparare a convivere con questo virus: i divieti erano necessari; per qualche parte lo saranno anche nei prossimi mesi, ma bisogna dare anche risposte politiche. Siccome il divieto è la risposta politica più semplice, bisogna iniziare a trovare delle risposte propositive; man mano bisognerà permettere le attività economiche prescrivendo severi protocolli di sicurezza. Se si continua con i semplici divieti, dopo la prima ondata della pandemia in primavera e la seconda ondata adesso a breve ci troveremo di fronte alla terza ondata, quella dei fallimenti e delle chiusure delle aziende; e poi di fronte alla quarta onda, quella della disoccupazione e della povertà. Dobbiamo puntare a costruire provvedimenti sempre più puntuali ed efficienti. Ad esempio il decreto ristori sta dando prove migliori sulla velocità di erogazione delle risorse rispetto ai primi provvedimenti, ma è stato meno efficiente nella definizione della platea dei beneficiari con tutto il discorso dei codici Ateco, quando invece l'unico principio dovrebbe essere quello della perdita del fatturato. Poi ci sono degli obiettivi più generali e di medio lungo termine da cui non dobbiamo mai distogliere lo sguardo, a cominciare dalla sostenibilità del nostro debito pubblico. il Governo fa un così grande affidamento sul *recovery fund* che con la legge di bilancio stima una retroazione fiscale positiva tanto da inserire queste risorse nei saldi di finanza pubblica. Come è stato detto in Commissione, è un elemento di rischio, anche perché le risorse vengono utilizzate per la copertura non di interventi straordinari, ma di politiche strutturali. L'Italia non può più permettersi di tornare a quella bassa crescita, ma per me il punto principale è un altro, ossia cosa accadrà all'Italia se, una volta terminata la fase di eccezionalità economica che vivremo con il *recovery fund*, questi progetti non saranno riusciti a determinare un cambio di passo nei livelli di crescita del Paese. È questa la partita che si gioca

debito, a quel punto, sarebbe un vero e proprio macigno per qualsiasi Governo e per qualsiasi politica, a prescindere dall'evoluzione del quadro europeo, ossia dell'interventismo o meno della BCE, della volontà o meno delle istituzioni europee di ritornare alla stagione di rigore finanziario. Quello che voglio dire è che noi con il *recovery fund* ci giochiamo la partita della vita. Per questo dobbiamo mettere in campo, col doveroso coinvolgimento del Parlamento e dei territori, delle Regioni e dei Comuni, un piano di progetti che siano all'altezza della sfida, che non disperdano le risorse in tanti interventi di piccolo e medio taglio senza alcun effetto moltiplicatore o di salto qualitativo del sistema. Anche perché nel frattempo ci sono altri Stati che hanno apparati burocratici molto più efficienti della nostra pubblica amministrazione. La mia prima preoccupazione, nel mettere in piedi le progettualità,

renderebbe il differenziale con gli altri Paesi incolmabile. Questo vale soprattutto, lasciatemelo dire, per la montagna che paga più di tutti il prezzo delle nuove restrizioni e su cui forse sarebbe utile aprire una riflessione

Per concludere, Presidente, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore dello scostamento di bilancio. Comprendiamo e sosteniamo il principio prudenziale che muove il Governo per via dell'incertezza sull'andamento pandemico. Allo stesso tempo, crediamo che sui progetti del *recovery fund* non ci sia più un minuto da perdere. Abbiamo apprezzato le linee di indirizzo. Adesso è giunto il momento della bozza di piano, con il doveroso confronto e coinvolgimento di Parlamento, Regioni Province e Comuni.

la sfida che abbiamo di fronte per l'Italia per i prossimi mesi è la crescita. È all'insegna di questo imperativo che dobbiamo programmare il nostro agire anche rispetto a come andremo a spendere le risorse che liberiamo attraverso lo scostamento di bilancio che ci apprestiamo a votare. Un voto, quello di oggi, che ci saremmo risparmiati volentieri ad un anno di distanza dall'inizio della pandemia perché sappiamo bene che scostamento di bilancio non significa altro che nuovo indebitamento. La bellezza di ulteriori 8 miliardi che vanno a sommarsi a quella montagna di debiti, 2.583 miliardi, che fanno del nostro debito pubblico il secondo più grande nello spazio europeo dopo la Grecia. In parole povere stiamo facendo un ulteriore brutto regalo ai nostri figli e ai nostri nipoti; continuiamo ad aggravare un'eredità che già oggi è salatissima per il Paese e per le giovani generazioni. Non si riesce però a fare diversamente dal momento che dobbiamo cercare di arginare quella drammatica crisi provocata dalla prima e, adesso, dalla seconda ondata di contagi da coronavirus, una crisi sanitaria ed economica di dimensioni disastrose. Ecco che, pur aumentando la spesa, è nostro dovere cercare almeno di contenere il danno facendo l'impossibile affinché il debito aggiuntivo che andiamo a produrre serva per lo più a finanziare investimenti e riforme strutturali, di modo che queste ingenti risorse possano andare, almeno in parte, a beneficio delle nuove generazioni, ad esempio, nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento di una società moderna, più vivibile, più sana e più attraente anche e proprio per i cittadini di domani. Ecco che è un bene che prevediamo una serie di misure a favore della genitorialità, della conciliazione tra mondo del lavoro e della famiglia indipendentemente dal genere. urgente infatti che in Italia si torni a mettere al mondo figli per garantire la tenuta del sistema pensionistico, ma anche per evitare la desertificazione umana in interi territori, nel Meridione d'Italia, come pure in zone appenniniche o periferiche. Il nostro Paese deve tornare ad essere un luogo a misura di bambino, cioè un Paese accogliente per tutti. Vanno nella direzione giusta anche le misure che abbiamo adottato a tutela dell'ambiente per favorire l'economia circolare e lo smaltimento dei rifiuti; misure capaci cioè di limitare l'impatto del cambiamento climatico e di rendere la nostra economia più sostenibile. Così come siamo ottimisti rispetto ai riscontri positivi che deriveranno dall'aver introdotto una forte decontribuzione per le assunzioni di giovani e di donne e che facciamo aiutando le aziende che hanno il coraggio di investire, sgravandole dal pagamento degli oneri previdenziali, cioè rendendo più convenienti le assunzioni di nuovo personale. Questo significa infatti creare opportunità per tanti giovani che da anni non avevano altre prospettive che l'emigrazione significa, al contempo, aiutare le imprese sane a ripartire per ricominciare a lavorare e guardare al futuro. La vera sfida da vincere, da qui ai prossimi anni, è la produttività; chiedere invece adesso la cancellazione del debito rischierebbe di essere controproducente perché vorrebbe dire trasmettere l'immagine di un Paese poco credibile. La strada per rimetterci in sesto è la ripresa economica e su questo bisogna investire. Dopo mesi nei quali nei successivi decreti abbiamo deliberato interventi miranti a far fronte all'emergenza, sempre di più iniziamo opportunamente a mettere in campo anche investimenti ed è urgente che sia così. La pandemia ci ha costretto ad intervenire con il più grande piano di spesa pubblica dal dopoguerra ad oggi, cercando di potenziare il sistema sanitario nazionale, creando posti di terapia intensiva, assumendo personale medico ed infermieristico e potenziando la ricerca sui vaccini. Abbiamo cercato poi di tamponare le situazioni di maggiori difficoltà economiche derivanti dal *lockdown*, con la proroga della cassa integrazione in deroga per tutti quei lavoratori che sono rimasti senza lavoro a causa della pandemia, con risorse a fondo perduto per coloro che hanno perso il proprio reddito a causa del Covid-19 e con il rinvio di adempimenti fiscali, pagamento di mutui, scadenze delle utenze. Insomma, una serie di misure volte a far fronte alla grave situazione provocata dal Covid-19, perché i mesi di *lockdown* hanno provocato effetti dirompenti sull'economia italiana, con un calo repentino attorno al 10 per e con un recupero che si presume sarà soltanto parziale l'anno prossimo, nella migliore delle ipotesi tra il 4 e 6 per cento. La pandemia, fra l'altro, purtroppo ha avuto conseguenze paralizzanti per interi settori produttivi, dal turismo alle attività ricettive alla ristorazione, anche a seguito della forte diminuzione dei flussi turistici verso l'Italia e anche il settore industriale è in sofferenza, anche a seguito della forte riduzione dell'*export* causata dal propagarsi del Covid anche in numerosi Paesi esteri. stessa cosa vale per il settore del commercio, che a sua volta ha subito una contrazione intorno al 21 per cento, anche a seguito del forte calo dei consumi. Con i provvedimenti che siamo andati via via a deliberare, come Italia Viva abbiamo insistito - e continuiamo a farlo - affinché si passi da aiuti emergenziali a misure che hanno un approccio diverso, di impulso alla ripresa e di investimento per il futuro. Penso alle misure di semplificazione volte a favorire la riapertura dei cantieri di infrastrutture pubbliche ma anche ai benefici fiscali che abbiamo introdotto per migliorare l'efficientamento energetico degli edifici, come pure alle risposte per l'innovazione digitale dell'intero Paese. Tutti incentivi dai quali sarà possibile ricavare grandi impulsi per l'economia. È su innovazioni di questo tipo che bisogna progressivamente puntare così da favorire un'accelerazione del processo di modernizzazione, intervenendo da subito anche su tutte quelle zavorre che per decenni sono riuscite ad imbrigliare l'Italia, a cominciare dalla burocrazia, dalla lentezza della giustizia, dalla fiscalità contorta, dalla farraginosità di parte della pubblica amministrazione. Bisogna puntare invece su investimenti che vadano a beneficio delle nuove generazioni e che contribuiscano a rendere più accogliente e più redditizio il nostro sistema. Solo così acquista un senso il nuovo scostamento di bilancio che ci apprestiamo a votare ed è di buon auspicio ed apprezziamo molto il fatto che Forza Italia e le opposizioni tutte, come da noi più volte auspicato, abbiano deciso di assumere un atteggiamento costruttivo, abbassando i toni e votando a favore dello scostamento di bilancio, perché la sfida è ardua ed affrontarla insieme ci aiuterà sicuramente a superarla meglio per il bene del Paese e dei nostri figli. Per questo ci auguriamo che il voto di oggi possa inaugurare una nuova stagione di dialogo e di maggiore collaborazione, in una fase storica così complicata, in cui si sente il bisogno di uno spirito di unità nazionale. Bisogna poi aggiungere, signor Presidente, che il fatto di doverci nuovamente indebitare per una cifra così elevata fa percepire quanto sia necessario ricorrere al MES, per una questione di costi innanzitutto, perché il MES è molto più conveniente di qualsiasi altra forma di credito. I buoni pluriennali del tesoro, con i quali finanziamo il nostro debito, ad esempio, hanno un costo di interessi molto maggiore.

il che fa sì che se utilizzassimo tutti i 36 miliardi di MES a disposizione potremmo risparmiare 370 milioni l'anno per un periodo di dieci anni, vale a dire che potremmo spendere complessivamente 3,7 miliardi di euro in meno, una cifra gigantesca, quasi la metà dello scostamento di bilancio che ci apprestiamo a votare tra poco. Cioè potremmo risparmiare metà del nuovo debito che andiamo a stilare oggi e nessuno capisce perché non dovremmo evitare questo spreco, visto che abbiamo già un debito pubblico così alto. In più, dovremmo ricorrere al MES anche per una questione di immediata disponibilità delle risorse, che potrebbero essere incamerate subito, invece i fondi del Next generation EU e degli altri programmi europei rischiano di essere disponibili solo con gravi ritardi a causa dei veti posti da Polonia ed Ungheria, come ci ha confermato appena stamattina il ministro Amendola. Questo significa che anche l'Italia dovrà aspettare a lungo per poter ricevere materialmente questi finanziamenti, cosa che non sarebbe necessaria se ricorressimo ai fondi previsti dal MES. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Governo, il tempo dei rinvii è finito, servono ingenti risorse. Il nostro sistema sanitario è nuovamente al collasso, c'è bisogno di medici, di infermieri, di terapie intensive, di telemedicina, c'è bisogno di fondi per mettere finalmente la parola fine alla pandemia e il MES può essere lo strumento più conveniente e più celere per provare a farlo. La situazione è troppo drammatica ed urgente per continuare ad opporre un no puramente ideologico, perché non solo siamo chiamati a spendere bene le risorse che riceviamo, ma abbiamo anche l'obbligo di spendere il meno possibile, visto che spendiamo sulle spalle dei nostri figli e dei nostri ragazzi. *(Applausi)*.

e non è la prima volta - a votare lo scostamento di bilancio. Non è la prima volta - lo dico con chiarezza noi votammo, in maniera responsabile, il primo e il secondo scostamento di bilancio, consentendo al Governo di utilizzare prima 20 miliardi e poi altri 55 miliardi.

è un nuovo debito, che tutti noi accendiamo mettendo una grave ipoteca sulla casa comune degli italiani. Abbiamo acconsentito a farlo, inizialmente per cifre imponenti, di fronte all'emergenza sanitaria ed economica. Ma al nostro atto di responsabilità non è seguito alcun atto del Governo, perché non avete poi mai corrisposto a quello che noi chiedevamo, cioè un confronto reale sugli emendamenti e, quindi, sulle norme legislative, su come sopperire, su come fronteggiare la crisi e su come creare i presupposti per la ripresa economica. Oggi torniamo non a darvi credibilità, perché questa credibilità - mi scusi, signor Vice Ministro - voi non l'avete più. Siete un po' come dei debitori insolventi, conclamati nella vostra insolvenza, perché oggi votiamo, corresponsabilmente, un altro scostamento di bilancio di 8 miliardi di euro, miliardi che si aggiungono ai precedenti, giungendo alla cifra di 108 miliardi di euro. euro. Oggi, in Aula, avete preso l'impegno specifico affinché questi 8 miliardi di euro siano destinati, in via quasi esclusiva o, comunque, prevalente, in aiuto a coloro che fino ad oggi hanno avuto poco o nulla, e cioè le imprese, le famiglie, i lavoratori autonomi, i titolari IVA, con una misura specifica e chiara, che è quella della sospensione dei pagamenti e del rinvio delle scadenze fiscali. Ebbene, questo vostro impegno noi vogliamo che sia specificamente mantenuto, tanto più che ci annunciate già che vi sarà un ulteriore scostamento di bilancio; e tanto più a fronte di quello che, purtroppo, sta accadendo con una manovra finanziaria che, in buona parte - come dicono la stessa Banca d'Italia, l'Ufficio di bilancio parlamentare e la Corte dei Conti

Noi ci aspettiamo che stavolta manteniate l'impegno, che andiate davvero in soccorso di chi sino ad oggi ha avuto poco o nulla, di coloro che sono i veri non garantiti in questo Paese, tanto più a fronte dei provvedimenti che hanno bloccato gran parte delle attività produttive,

e il numero di occupati si riduce: riducendosi la base produttiva e chiudendo le imprese, si chiudono anche i contratti di lavoro, oltre quelli che non sono stati rinnovati per le follie del decreto dignità. Parliamo di un milione di occupati in meno. Ebbene, a fronte di questa situazione davvero difficile e drammatica, non basta avere risorse in debito, che comunque poi dovranno essere ripagate,

e con un indebitamento di quasi 2.600 miliardi. Quindi meno produzione, meno occupazione, meno prodotto interno lordo e più debito pubblico: rischiamo davvero il collasso finanziario e sociale del Paese. È necessario, quindi, che ci sia una svolta che ancora voi non realizzate, a fronte di un'Europa che - a differenza di quello che la sinistra poco fa propagandava in questa Aula è sì cambiata, ma non nella direzione che voi volevate, bensì appunto nella direzione che noi chiedevamo ancor prima della crisi. crisi. L'Europa cambia quando, a fronte della drammaticità della situazione, si rende conto finalmente di quello che noi dicevamo prima addirittura in una situazione che non era quella attuale - e cioè che occorreva rivedere il Patto di stabilità. Non lo dicevate voi: lo dicevamo noi. L'Europa ha addirittura sospeso il Patto di stabilità e tale sospensione è stata prorogata di un altro anno; abbiamo due anni di tempo

e condivide il debito pubblico. Persino esponenti della maggioranza cominciano a parlare della necessità di cancellare il debito pubblico. Persino un Presidente del Consiglio di questo Paese, un europeista che studia e lavora a Parigi, Enrico Letta, ci dice

E lui stesso dice di prendere il denaro del MES, che nessuno sta attivando, e di utilizzarlo direttamente attraverso la Commissione europea, perché altrimenti li è congelato e resterà congelato. Siete voi che fate un dibattito ideologico sul MES. Persino alcuni Presidenti del Consiglio di questo Paese, più avveduti, vi dicono di finirla con questa storia, che è una bandiera inutile, una falsa bandiera, e di andare a prendere le risorse dove ci sono e soprattutto di utilizzarle dove davvero servono.

Torno alle origini: siamo stati noi a chiedervi di fare uno scostamento di bilancio significativo nel primo provvedimento, perché ricordo a tutti che voi non avevate capito la drammaticità della situazione e avevate portato un provvedimento da una manciata di miliardi. Soltanto di fronte alle richieste delle opposizioni e di Fratelli d'Italia quel provvedimento ha preso consistenza, con 20 miliardi di indebitamento. di indebitamento. Capite le cose sempre con estremo ritardo, perché siete lontani e in ritardo rispetto alla realtà del Paese. Spero che stavolta, di fronte al nostro ennesimo atto di responsabilità, vi sediate davvero a discutere, con una visione del Paese, su come indirizzare le risorse che comunque ci sono. Le risorse infatti ci sono, sia come indebitamento, grazie all'iniziativa

la crescita non si produce per decreto - lo sappiamo tutti - ma può essere bloccata per decreto e voi avete fatto una serie di misure che hanno impedito la crescita. vogliamo che si facciano le misure che possano consentire al Paese di riprendere a crescere con fiducia. Diamo certamente fiducia al Paese, non al Governo, con questo scostamento di bilancio che significa debito sulle spalle di tutti e che noi vorremmo

facciamo un passo in avanti rispetto alla situazione precedente. È vero che sono stati votati dalle opposizioni anche i primi due scostamenti -

né di un inciucio, né tantomeno del tentativo di confondere il ruolo tra maggioranza e opposizione, finalmente - dico finalmente, perché l'ho sostenuto

e si comincia forse a lavorare insieme. Lo si fa, colleghe e colleghi, per dare una prospettiva e un futuro al nostro Paese, ferme restando le diverse posizioni politiche; per dire ai cittadini italiani che questo Paese ha una prospettiva nel cambiamento e nell'innovazione. Con questo scostamento daremo una risposta alle piccole e medie imprese, all'Italia di partite IVA e ai professionisti. Non condivido la narrazione per cui negli ultimi mesi verso questi soggetti non è stato fatto nulla. Sapete anche voi che non è vero: è una narrazione sbagliata. Tuttavia, è certamente questo uno dei punti più delicati e critici della crisi economica e sociale che stiamo vivendo. E penso che, dopo i rinvii delle scadenze dell'IVA, dei contributi previdenziali e dell'IRPEF - fondamentali visto che la prima scadenza sarebbe

dobbiamo costruire una strategia vera in grado di lavorare sulla riduzione dei fatturati,

e fare un'operazione di equità e trasparenza. Anzi, spero che sarà possibile allora poter verificare e prestare attenzione

in un sistema del lavoro che ha bisogno di una riforma radicale. Detto questo, vorrei vorrei chiarire altri due punti. Dobbiamo anzitutto sconfiggere la pandemia. Mettiamoci d'accordo su un elemento che credo sia oggettivo: sconfiggere la pandemia è una priorità per la salute dei cittadini, tanto quanto per l'economia. Se la pandemia continua, l'economia non ha ripresa. ripresa. Spero che dopo queste settimane si sia chiusa definitivamente la discussione sulle norme da utilizzare. Il Covid c'è

che sia in grado di garantire la gestione fino all'arrivo dei vaccini. Non possiamo certo dimenticarci di agosto

superando anche i limiti che abbiamo avuto in questi mesi sui trasporti, sulle soluzioni alternative in tema di aule e su un nuovo piano regolatore degli orari

di bilancio, per favore, superiamo tutti i vincoli nell'ambito delle assunzioni di personale in sanità.

sia capace di gestire i grandi investimenti per dare produttività e qualità alla crescita, una qualità sociale ed ambientale,

quando parliamo di bambini o di anziani non parliamo di frigoriferi o di televisioni; ci vuole, quindi, un sistema di accreditamento

Questa è la vera sfida della riforma del *welfare,* e non il dibattito vecchio e inconcludente tra pubblico e privato. Abbiamo tanto da fare, ma credo

rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, quello che ci apprestiamo a votare è il quinto scostamento di bilancio dall'inizio della crisi. Ormai votiamo scostamenti quasi con la stessa consuetudine con cui votiamo il calendario sui giornali se ne parla più per i numeri dei voti al Senato che per quelli di finanza pubblica. Sulle nostre caselle di posta elettronica non arrivano le proposte e le sollecitazioni di cittadini e parti sociali che accompagnano altri provvedimenti. Sembra quasi di trovarsi di fronte a un atto dovuto, a un passaggio formale e burocratico piuttosto che sostanziale. È abbastanza incredibile se solo pensiamo che il tema del debito pubblico e degli equilibri di finanza pubblica ha rappresentato la pietra angolare della politica economica in Italia e in Europa negli ultimi decenni. Altri Governi e altri Parlamenti si sono mossi nel sentiero stretto degli "zero virgola" per provare a contemperare crescita e risanamento finanziario. La crisi pandemica ha cambiato tutto ed è giusto che sia così, ma questo non ci esime dal considerare tutte le implicazioni delle scelte che stiamo prendendo, tutti i rischi che si riproporranno una volta usciti dalla pandemia se non accompagniamo le scelte di bilancio con altre scelte politiche: in sintesi, se non usiamo bene lo spazio fiscale che stiamo aprendo. Anche il voto favorevole delle opposizioni allo scostamento in esame è un fatto molto positivo, che ci consente di passare dai numeri sbagliati (i margini parlamentari) ai temi giusti (come spendere presto e bene le risorse che stiamo mobilitando). Rispetto alla crisi finanziaria del debito del periodo 2008-2011, l'Unione europea si sta muovendo nella direzione giusta. Alcuni errori di allora sono stati compresi e la Commissione ha subito sospeso il Patto di stabilità e si sta avviando, non senza difficoltà ma con una forte ambizione di fondo, il piano Next generation EU per una risposta incisiva e condivisa alla crisi. Come ci ha spiegato lo stracitato Mario Draghi, è il momento del debito buono, anche se noi italiani - ci aiuterebbe ammetterlo - in passato siamo stati maestri anche di debito cattivo per ragioni elettoralistiche piuttosto che di crescita e di giustizia sociale. Ora però i bilanci pubblici devono ripianare i debiti privati, che altrimenti strozzerebbero famiglie e imprese, affossando le nostre economie. Anche il debito buono, tuttavia, avrà effetti politici ed economici nel futuro, non perché dobbiamo restituirlo alla scadenza, come capita a famiglie e imprese - il debito pubblico è diverso da quello privato - ma perché il debito pubblico incide sulle scelte che Governi, imprese e famiglie potranno fare in futuro. Usando giustamente la nostra sovranità oggi per uscire dalla crisi, stiamo ponendo vincoli sulla nostra sovranità domani, su ciò che potremmo fare dopo la pandemia per dare risposte ai cittadini e dobbiamo esserne consapevoli. È il momento del coraggio delle scelte, ma il coraggio richiede senso di responsabilità, altrimenti diventa qualcos'altro. La risposta ai debiti che stiamo contraendo oggi sarà una sola, se ci sarà. E non penso alla crescita economica, anche se, certo, senza crescita non c'è sostenibilità del debito. La crescita, però, è una condizione necessaria e non sufficiente per la sostenibilità del debito. Da sola non basterà. La risposta che serve è più Europa, più crescita e più Europa. Servono entrambe: una sola di queste due cose per noi rischierebbe di non essere sufficiente e le due cose si tengono tra loro. loro. Solo se useremo bene le risorse che l'Europa ci sta per mettere a disposizione, saremo credibili nel chiedere un salto di qualità nella costruzione europea, che serve a tutti gli Stati membri e non solo all'Italia. E solo se l'Europa diventerà una vera unione fiscale, che completi quella commerciale e quella monetaria, le nostre leggi di bilancio e le nostre riforme potranno trovare lo slancio necessario per agganciare una crescita sostenuta e sostenibile. Più crescita e più Europa servono entrambe ed entrambe si tengono tra loro. Prendiamo il tema mediatico della cancellazione dei debiti dovuti al Covid. Non è il momento dei conservatorismi. Dobbiamo pensare a ciò che sembrava impensabile poco tempo fa. Così come la politica monetaria sta usando strumenti eccezionali, anche quella fiscale può disegnare strumenti eccezionali di fronte all'eccezionalità della crisi che stiamo vivendo, ma pensare l'impensabile non può esimerci dal pensare. A maggior ragione, quando si avanzano proposte eccezionali, dobbiamo pensare a tutte le conseguenze economiche e politiche che comportano. Gli *slogan* e gli appelli non bastano. Non dobbiamo parlare - per esempio - di cancellazione perché, a differenza dei debiti tra Stati o verso organizzazioni internazionali come nel caso di quelli di molti Paesi in via di sviluppo - parliamo di debiti detenuti in gran parte da investitori istituzionali e famiglie, e penso che nessuno voglia cancellarli per fare *default* a livello europeo o italiano. Dobbiamo parlare, casomai, di sterilizzazione monetaria o di mutualizzazione fiscale dei debiti da Covid. Se vogliamo parlare di entrambe le cose (sterilizzazione monetaria e mutualizzazione dei debiti), si richiedono scelte enormi e difficili. Una parziale monetizzazione dei debiti richiede una modifica dei trattati europei e del mandato della Banca centrale, preservandone l'autonomia, e sottolineo quest'ultimo aspetto. Una parziale mutualizzazione dei debiti richiede una vera unione fiscale che completi l'unione monetaria con un'autorità politica non tecnocratica, che sposti a livello europeo un pezzo delle nostre tasse e dei nostri debiti.

non ne esce l'Italia perché, con il nostro debito, avremo un fardello i cui costi prima o poi diventeranno una zavorra insostenibile. Per questo le risposte ai debiti che stiamo contraendo oggi non arriveranno da *slogan*, da appelli o da alchimie finanziarie: possono arrivare solo dalla conferenza sull'Europa e da una nuova idea di Europa. Il momento è ora, perché in politica le fasi due non esistono quasi mai, se non nei sogni o nelle ipocrisie di chi le invoca. È nel mezzo di una crisi come quella che abbiamo di fronte che dobbiamo rilanciare la costruzione europea o non riusciremo a farlo domani. L'Italia deve mettersi alla testa di questa battaglia per una nuova sovranità fiscale europea. E deve farlo innanzitutto con la credibilità che solo un piano nazionale per la ripresa e per la resilienza serio, attuabile e basato su priorità chiare, potrà darci, non per le condizioni che ci chiede qualche burocrate, ma per le scelte che vogliamo fare noi, come italiani, di fronte alle crisi e alle ingiustizie sociali di questo Paese.

e le speranze di milioni di giovani, che abbiamo lasciato troppo soli a sostenere il costo della crisi, senza investire sulle loro opportunità, sulla loro formazione, sulla garanzia del loro reddito in ingresso nel mondo del lavoro, in un momento così drammatico. drammatico. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico alla relazione presentata dal Governo, ribadisco che questo voto è non un atto formale o un passaggio burocratico, ma una scelta da noi vissuta con consapevolezza e responsabilità, rispetto a tutto quello che comporta. Consapevolezza e responsabilità da domani, metteremo nelle sfide enormi che si aprono: spendere bene le risorse italiane ed europee che stiamo mobilitando e costruire un'Europa fiscale e politica, che completi l'unione commerciale e monetaria, per raggiungere obiettivi di crescita, di giustizia sociale e di sostenibilità del debito, per tutti noi e, non da ultimo, per le future generazioni di italiani e di europei.

Signor Presidente, onorevole Vice Ministro, colleghe e colleghi, l'Italia è purtroppo ancora investita dalla pandemia da Covid-19,

Servivano reazioni tempestive e programmazione dei rischi. Fin dall'inizio si parlava di seconda fase e di seconda ondata e già ora si parla purtroppo anche di terza ondata. L'onorevole Vice Ministro è qui per chiedere, a nome del Governo, il voto sul quarto scostamento di bilancio per 8 miliardi di euro. Non ci siamo mai opposti alle precedenti richieste sullo scostamento di bilancio,

abbiamo fatto delle proposte, che il Governo non ha ascoltato: non vi siete confrontati e non avete discusso alcunché. Vi siete limitati a rincorrere il passato, con chiusure disordinate e di non facile comprensione - almeno per gli italiani

Signori del Governo, comprendiamo le difficoltà. Non comprendiamo però il timore di affrontare le questioni. Non comprendiamo l'incapacità - al momento totale - di avere un disegno di respiro, di avere il coraggio di pensare e sfidare il futuro, pensare al dopo anche. Ed è questo che chiediamo. Sappiamo che l'economia del dopo sarà diversa, e lo sarà per tante ragioni: per il cambiamento tecnologico, per le abitudini che sono cambiate - comunque un impulso al cambiamento delle abitudini c'è per una serie di processi di impresa che hanno subito un mutamento, che probabilmente sarà anche più accentuato. Va accompagnato e va regolato, e lo Stato ha bisogno di entrate e non di soli debiti. Lo diciamo responsabilmente: lo Stato ha bisogno di entrate e non solo di debiti. Ecco perché vi diciamo - e lo facciamo nell'interesse degli italiani - come ha fatto il nostro presidente Berlusconi qualche giorno fa,

decreto-legge ristori 4 da 8 miliardi, preannunciando fin d'ora che ci sarà un ristori 5, quindi con valutazioni che faremo successivamente. Le proposte di Forza Italia, in gran parte confluite nella risoluzione unitaria del centrodestra - e ringrazio i colleghi di Lega e Fratelli d'Italia - dicono basta alla confusione. *(Applausi).* Basta con la confusione: serve anzitutto un semestre bianco. Basta con elemosine a pioggia: servono ristori con riferimento ai costi fissi. *(Applausi);* ristori a tutte le attività economiche, e quindi in base al fatturato e - come detto - alla parte dei costi fissi rapportati.

non tutto si può ristorare; si può però dare tranquillità e meno angoscia dimostrando che lo Stato c'è ed è al fianco dei propri cittadini. Il semestre bianco chiesto dal nostro Presidente è anche questo.

chiediamo di non tartassare ulteriormente con sanzioni e pene pecuniarie coloro che hanno dichiarato e, quindi non sono evasori, ma non sono in grado - viste le entrate - di far fronte ai loro impegni. Oggi Forza Italia, su indicazione del presidente Berlusconi, unitamente ai colleghi di centrodestra, è qui: critica ma propone; è qui a valutare lo scostamento e a votarlo, perché quando si è in guerra non ci si distingue per colore.

risoluzione proposta dalla maggioranza sullo scostamento di bilancio.

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, facciamo un rapido riassunto delle puntate precedenti.

Stiamo per votarne - se questa è una notizia, ve la do - uno da 8 miliardi di euro e già sappiamo che ne arriverà uno da 20 miliardi. Questo lo dico per chi, fuori dai palazzi, non sapesse come stanno andando le cose. Già da questo si evince che nella strategia del Governo l'approccio è stato quantomeno frammentario. Da questi banchi qualcuno a marzo vi chiese di riflettere sul titolo di un libro non sprecare una crisi come questa; la richiesta implicita era di intervenire in modo incisivo e tempestivo. Questo non è successo, ma è il passato. ma è il passato. Guardiamo al presente e vediamo se si può osservare un'evoluzione. Un'evoluzione positiva la notiamo nell'atteggiamento del Governo. Abbiamo visto in questa maggioranza che finalmente si comincia a vedere qualcosa che va, ma resta ancora molto che non va. Io comincerò dal sottolineare quello che va. Si nota una certa resipiscenza, finalmente; si nota un inizio di ascolto. Entrano finalmente nel radar di questo Governo gli autonomi, i professionisti. *(Applausi).* Quando ho letto «autonomi» nel testo ho pensato che fosse un attacco di nostalgia canaglia, poi invece, quando ho visto accanto la parola «lavoratori», ho capito che si parlava effettivamente di non tutelati, che finora questo Governo aveva un pochino lasciato da parte e qualche volta direi anche bullizzato con i meccanismi del *click day*. Di questo si fa atto di ammenda, e ci sono tanti buoni propositi nel testo di maggioranza, indubbiamente. Si è anche capita un'altra cosa: che l'attesa del *lockdown* è essa stessa il *lockdown*, e che quindi fare tanta differenza fra codici Ateco e fra zone in un momento in cui il pessimismo e anche l'incertezza - va detto, non se la prendano a male gli onorevoli membri del Governo - sparsa a piene mani da questo Governo,

questo lo considero un dato positivo e significa dal punto di vista politico una cosa: il centrodestra unito fa paura a una maggioranza divisa. *(Applausi).* Ringrazio i colleghi di centrodestra con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi giorni per addivenire a una posizione unitaria, che però congiunzione avversativa - è stata ripresa solo in parte dal Governo, nonostante tutta una serie di profferte iniziali. Molte cose sono rimaste fuori e per chiarire il motivo per il quale, invece, le si sarebbe dovute tenere dentro vorrei fare una breve riflessione. Vede, signor Presidente, nel Medioevo analogico - quello che tutti ricordiamo la politica distributiva veniva fatta da Robin Hood, che usava le sue frecce per rubare ai ricchi e dare così dire, una rudimentale politica redistributiva che in qualche modo combatteva, in un mondo meno complesso di quello odierno, la disuguaglianza che era molto più accentuata - per ora - rispetto ad oggi. oggi. In questa diversa temperie culturale i fautori, i propugnatori del futuro Medioevo digitale, quello della decrescita felice, armati di frecciatine verso i nostri colleghi di centrodestra, citano qui in Aula Saez e Zucman, ma io aggiungerei anche il loro sodale Piketty, che ci dice nel XXI secolo

di sinistra che oggi siede su questi banchi, e vi chiarisco un concetto, rivolgendomi innanzitutto al collega Nannicini, che per *standing*, per posizione accademica, forse il problema della disuguaglianza non va risolto a valle con interventi fiscali, ma a monte sul mercato del lavoro ed è proprio in questo che l'Europa non ci aiuta e qui qualcuno lo sa, anche se fa finta di non saperlo. saperlo. Il mondo della svalutazione interna, infatti, il mondo della compressione dei salari come unica risposta agli *shock* macroeconomici è il mondo della disuguaglianza: ma questo mondo va bene, perché ci viene raccontato che la crisi ha cambiato tutto ed è giusto che sia così. così. Insomma, è giusto mica tanto: riflettiamo un attimo su ciò cui stiamo assistendo. Stiamo assistendo ad una confessione: il fatto che delle regole fiscali, di cui da sempre gli economisti conoscono l'assurdità, vengano disapplicate adesso che nei guai sono i Paesi del Nord significa una cosa sola: per questa Europa che a voi piace tanto un bambino greco conta meno di un bambino tedesco *(Applausi)* e voi, nel difendere questo progetto, ve ne rendete complici, mentre andate in giro a dare a vanvera del negazionista a destra e a sinistra a chi esercita un diritto di critica e vi associate a questo nuovo nazismo. Questo non è molto carino da parte vostra, soprattutto da parte di quelli che in quest'Aula siedono là di fronte a me.

senza ovviamente nulla togliere alla funzione redistributiva del sistema fiscale, esiste una radice del problema molto evidente - ragioniamo un attimo sulle tante proposte che in una lunga giornata e mezza di trattative e di negoziato sono cadute per non essere state riprese dall'attuale maggioranza e dal Ministero. ad esempio, cui credo coralmente teniamo nel centrodestra, era quella di portare avanti finalmente un ammortizzatore sociale unico per semplificare la vita dei lavoratori *(Applausi)* e, se permettete, anche dei consulenti del lavoro

naturalmente altri interventi che, a nostro avviso, sarebbero stati opportuni. È venuto il momento delle circostanze eccezionali e dei grandi passi. Guardate, c'è un intervento, il primo che mi sono sentito raccontare dal Consiglio

noi condanniamo i nostri imprenditori migliori ad andarsene e poi piangiamo sul latte versato. C'erano però anche altre proposte. un certo odio ideologico verso il ricco, verso i tanti sceriffi di Nottingham che voi vedete in giro, ma che in Italia non ci sono, anima questa maggioranza o pezzi di essa, perché essa è molto variegata. Noi avevamo anche, fin da luglio, proposto un intervento serio sull'IMU. L'intervento che l'aveva alzata ha fatto diminuire, secondo il Centro studi di Confedilizia, i valori immobiliari del 27 per cento. Che senso ha però questa distruzione di ricchezza? A chi fa del bene? Neanche al gettito, neanche all'erario. Lo stesso vale peraltro per la distruzione di ricchezza causata dal *bail-in* e da tutte queste altre belle cose europee, che a voi piacciono tanto. Bene, io vi ho detto che c'è ancora strada da fare se gli intenti mostrati in questa risoluzione sono effettivamente sinceri e si tradurranno effettivamente da impegni in gesti concreti

del fatto che l'unico investimento produttivo è quello in capitale fisico. Tanti colleghi, anche accademici, si riempiono la bocca di capitale umano, poi vengono qui in Aula a chiamare «spreco» la spesa per infermieri, poliziotti e vigili del fuoco.

Signor Presidente, Governo, colleghi, qualche mese fa Alfonso indossa di nuovo la divisa, torna sull'ambulanza e con i suoi vecchi colleghi ricomincia a correre per salvare vite. Durante i soccorsi però si contagia e in pochi giorni finisce in terapia intensiva, dove viene intubato e poi muore. Questa è la storia di Alfonso Durante, infermiere in pensione tornato sull'ambulanza a combattere il virus Come Alfonso, ci sono tanti operatori sanitari che stanno dando il meglio di sé, la propria stessa vita per salvare quella degli altri. Grazie Alfonso e grazie a tutti quelli che stanno combattendo questa battaglia in prima linea. Questo tempo sospeso è carico di storie, ognuno di noi sta scrivendo la storia e la scelta di quale personaggio interpretare spetta solo ed unicamente a ciascuno di noi. Ci sono le storie degli insegnanti che per mantenere alta l'attenzione dei propri studenti durante la didattica a distanza hanno creato moduli di studio fantasiosi e geniali, come Sandro Marenco un professore di inglese e tedesco in un liceo scientifico di Alessandria che, per non lasciare soli gli studenti d'estate e per stimolarli ad approfondire le materie, ha creato l'*hashtag* «ripassiamo insieme», diventato virale. Ci sono le storie degli imprenditori che hanno saputo riconvertire le proprie aziende e valorizzare il personale dipendente per non fargli perdere il lavoro. Grazie a tutti questi docenti, a questi imprenditori e a tutti coloro che hanno saputo immaginare un mondo nuovo. Erano decenni infatti che si parlava di digitalizzazione e *smart* *working*, ma fino ad oggi sembravano utopie, mentre adesso sono realtà. Oggi lavoratori, insegnanti e studenti vivono e operano in un unico spazio che si chiama infosfera.

ha dimostrato che per il 41 per cento degli intervistati passando allo *smart working* l'efficacia lavorativa è migliorata e per un altro 41 per cento è rimasta identica; ha dimostrato inoltre che il 56 per cento dei lavoratori ha approfittato del periodo di *lockdown* per dedicare una parte del tempo alla formazione per migliorare le proprie competenze digitali, la conoscenza del codice degli appalti e dell'anticorruzione. Lavorare da casa quindi non ha significato smettere di lavorare, né lavorare meno. Abbiamo affrontato per primi in Europa questa pandemia e tutto il mondo, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità, ha riconosciuto il merito dei provvedimenti messi in campo da questo Governo. Abbiamo seguito il metodo scientifico attraverso il monitoraggio, l'analisi dei dati utilizzando numerosi parametri, l'attuazione di misure graduali, adeguate e modificate in base all'andamento della pandemia e alla tenuta del nostro tessuto economico. In pochi mesi abbiamo stanziato risorse per l'equivalente di tre manovre finanziarie. Con i decreti cura Italia e rilancio abbiamo investito 75 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana, 8 miliardi per rimettere in piedi la nostra sanità (depotenziata e destrutturata da decenni di tagli), 28 miliardi di aiuti alle famiglie, 15 miliardi per la cassa integrazione, 8 miliardi per autonomi e partite IVA, 3,5 miliardi per congedi parentali e *voucher* per nuclei famigliari, 18 miliardi per le imprese (di cui sei per i contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese), quattro miliardi per cancellare il saldo 2019 e l'acconto 2020 IRAP, 2,5 miliardi per il credito d'imposta e la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, 6 miliardi per i Comuni e gli enti territoriali, un miliardo per il reddito di emergenza. Adesso, con i decreti ristori, stiamo dando ossigeno alle attività che hanno subito danni per le chiusure delle zone rosse e per consentire ai Comuni di adottare ulteriori misure urgenti di solidarietà.

Ci saranno ulteriori difficoltà, tutti ne siamo amaramente consapevoli e pensiamo con preoccupazione alle tante attività legate al turismo invernale che non potranno riaprire e per le quali vanno messe in campo norme di sostegno urgenti. Ci avviciniamo inoltre alle festività natalizie, che richiamano alla nostra mente l'immagine di famiglie riunite, di serate tra amici, di abbracci. Non dobbiamo però dimenticare un'altra immagine, quella di una figlia in piedi sul tettuccio della propria auto parcheggiata accanto alla finestra della stanza di ospedale in cui è ricoverata sua madre e che dal tettuccio muove le braccia ben sapendo di non essere vista, ma certa di riuscire a trasmettere il suo amore a chi sta lottando per sopravvivere a pochi metri da lì. Oggi sembra impossibile trovare una via d'uscita che accontenti tutti. Come si conciliano esigenze così distanti? Voglio raccontarvi una storia, anche per smorzare un po' i toni di questa discussione. Tanto tempo fa in Medio Oriente viveva un uomo che alla sua morte lasciò ai suoi tre figli 17 cammelli in eredità. Ad uno ne donò la metà, al secondo un terzo, al più giovane un nono. Questi ragazzi provarono per mesi a dividere l'eredità secondo la volontà del padre, ma non ci riuscirono, perché 17 non è divisibile per 6, non è divisibile per 3 e così chiesero aiuto ad una saggia, che dopo aver ragionato a lungo propose loro una soluzione: donò loro il suo cammello, in modo che ne avessero 18 e non più 17. Così il calcolo diventò più semplice:

La somma però di 9 più 6 più 2 è proprio 17 e quindi i ragazzi restituirono alla donna il diciottesimo cammello. Questo per dire che spesso le nostre posizioni sembrano davvero inconciliabili le difficoltà insormontabili. In questo momento, le risorse ci appaiono certamente limitate per essere distribuite equamente e risolvere i problemi esistenti. Eppure, a volte basta solo cambiare prospettiva: in fondo, siamo una grande famiglia. L'umanità è una grande famiglia. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è raggiungere il bene comune. Oggi siamo felici che le opposizioni abbiano accolto il nostro invito a collaborare per il bene dei cittadini, perché solo insieme possiamo dare una mano a tutti quelli che, in questo momento, hanno paura di non farcela: a chi teme di aver perso tutto, a chi vede avvicinarsi l'ombra della depressione, a chi ha perso i propri cari o il proprio lavoro. Di notte, le ansie, le paure, il dolore diventano più forti, ma appena sorgerà il sole ci sentiremo di nuovo padroni del nostro tempo. Non sappiamo quando tutto questo sarà finito, ma sappiamo per certo che quel giorno arriverà. Siamo consapevoli che lo scostamento di bilancio che votiamo oggi è un ennesimo piccolo passo per raggiungere il traguardo della ripresa economica di questo Paese siamo anche certi che ci aspetta ancora un grande e duro lavoro, ma ne usciremo più forti solo se tutti sapremo operare insieme, uniti per il bene comune, mettendo in gioco la parte migliore di noi stessi. Oggi parliamo di 8 miliardi di euro, che serviranno per finanziare i nuovi decreti ristori. Dobbiamo continuare a sostenere le imprese e i lavoratori che si trovano in difficoltà nelle zone più ad alto rischio e, quindi, soggetti a più chiusure. Con queste nuove risorse intendiamo congelare tutta una serie di proroghe fiscali, che consentiranno al tessuto economico e produttivo di affrontare con più serenità i prossimi mesi. Ed è con questa consapevolezza che oggi il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questa misura, richiesta e necessaria per fronteggiare la recrudescenza della pandemia e supportare imprese e famiglie.

come possiamo credere davvero ad un Governo che apre, che allarga, che condivide, quando poi lo stesso Governo si restringe e si appoggia ad un Arcuri supercommissario: all'emergenza Covid-19, alla gestione del piano vaccinale e persino all'Ilva? Affidate ad un uomo solo emergenze che, prese singolarmente, farebbero perdere il sonno a chiunque. Evidentemente, o Arcuri è paranormale o voi siete scarsi; oppure non c'è nessun emergenza da gestire, se un solo uomo ne deve gestire tre. Il problema non è lo scostamento di bilancio, ma il vostro scollamento dagli italiani e il vostro scollamento da questioni troppo più grandi di voi. Voi siete abituati alla metaforica genuflessione. Ora al sistema Benetton (vero, Patuanelli?), ora a Big Pharma (vero, Speranza?), ora al condannato Alessandro Profumo (vero, Gualtieri?). Qui manca la visione. Altro che dare i soldi alle partite IVA: 5 miliardi alle banche sono soldi. E poi ho letto su «La Verità»: 72 milioni di euro dati come provvigione per le mascherine, tanto che è partita una segnalazione in Banca d'Italia dall'Antiriciclaggio. Quelli sono soldi. I problemi sono più grandi di voi. Che ne sapete del dramma delle famiglie, dove i genitori, se perdono il lavoro a cinquant'anni, diventano fantasmi? Effetto Covid-19: a rischio povertà altri due milioni di famiglie. Vi riparate dietro il reddito di cittadinanza, salvo poi lasciare per strada i *navigator*, ma non Mimmo Parisi, perché è amico vostro. Come se la sfida fosse solo assistere e non il rilancio dell'occupazione e dei salari; ma è la piena occupazione ad essere la grande sfida della classe dirigente. Voi parlate dei decreti ristori, evidentemente poca cosa se la mafia acquista spazi e potere. I vostri decreti sono sempre due passi indietro rispetto alle esigenze (il turismo invernale, lo vedremo con il prossimo scostamento). Le bollette sono fatte così: ben oltre il 60 per cento sono composte dagli oneri di sistema. Ma non vi vergognate? È in corso un'apocalisse del commercio e non la vedete. Quasi 100.000 i fallimenti in sei mesi. Da aprile a settembre sono cessate 98.000 imprese. La filiera della moda sta collassando perché vi sfuggono le logiche sia della filiera produttiva sia della catena dei pagamenti. I titoli di credito a scadenza di chi ha comprato la merce diventeranno incaglio e gli avvisi bonari diventeranno cartelle esattoriali. Se non rivedete le regole della centrale rischi, l'economia reale vi scoppierà in faccia. È inutile che prorogate le scadenze delle tasse; che vi piaccia o no, siete costretti a un *reset* fiscale concordato oppure lo sciopero fiscale sarà l'autodifesa del commercio. E, di fronte a uno Stato che non paga, nessuna lezioncina di rispetto delle regole varrà, perché i primi a non pagare siete voi, quindi siete disonesti. di fronte a un Governo che nomina nelle partecipate di Stato gli imputati, che non rimuove gli amministratori delegati condannati, che tratta con i *manager* che da lì a poco saranno arrestati o che regala soldi alle banche per coprire il sistema relazionale, di cosa ci sorprendiamo? Altro che scostamento di bilancio; scostatevi voi, perché la situazione si sta facendo pesante e non avete il *curriculum* per affrontarla.

Signor Presidente, molto più pacatamente, io rispetto ovviamente il terreno dell'intesa, anche se non mi è chiaro. Oggi pomeriggio ho ascoltato con grande attenzione questo dibattito e mi sono perso tra Robin Hood e lo sceriffo di Nottingham; non ho capito su cosa si è costruita l'intesa, se non una serie di insulti dei colleghi dei 5 Stelle verso Forza Italia. Quello che capisco - ed è per questo che Azione e Più Europa si asterranno nel voto di oggi che sui ristori alle imprese ci sono le idee così chiare che, mentre il Parlamento sta convertendo il primo decreto-legge ristori, è stato scritto il secondo, ideato il terzo e pensato il *quater*. Devo dire che questo è il modo migliore per lasciare indietro costantemente segmenti dell'economia, categorie, settori produttivi, per una risposta che ha tutto tranne l'organicità. Sui temi della sanità ho ascoltato con grande attenzione e anche grande rispetto la narrazione anzi oggi potremmo chiamare il "ristori telling") sui temi degli operatori, ai quali va tutta la nostra solidarietà. Ma, se volete aiutare la sanità metteteci i soldi; e sapete dove andarli a trovare. L'ultimo punto: non ci sottrarremo mai - lo dico al Governo - da una disponibilità vera alla collaborazione fatta sui provvedimenti. Chiamateci a deliberare, decidere, legiferare sulle borse di specializzazione in medicina, sul piano Amaldi sulla ricerca universitaria e su una reintroduzione vera di Industria 4.0. Voi oggi avete rimesso il titolo, ma non avete finanziato i *competence center* e non avete finanziato gli ITS. Queste sono le battaglie che Più Europa e Azione faranno in questo Parlamento, perché, se le intese nascono come oggi si è sviluppato questo dibattito, credo che per il Paese non sia una buona notizia.

della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione. Ricordo che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.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

secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Voglio iniziare il mio breve intervento citando Maria Montessori: «Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo». È nostro dovere ribadire con forza la necessità del rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza, dei bambini e degli adolescenti prima di tutto come persone e uomini di domani. Occorre affermare con forza che i bambini vengono prima di tutto e di tutti e non devono essere discriminati promuovere la frequenza scolastica, contrastando in tutti i modi il fenomeno, ancora purtroppo diffuso, dell'abbandono scolastico. Non si potrà e non si dovrà mai affermare che alcuni bambini hanno meno diritto di altri, solo perché meno fortunati. Penso in questo caso ai bambini con disabilità, ai bambini fragili o che vivono in condizioni ambientali molto disagiate. Ciononostante, ancora oggi, molti di loro, anche in Italia, sono vittime di violenza o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di disagio sociale ed isolamento. Non possiamo dimenticare i tanti bambini del mondo che muoiono ancora di fame e di stenti o sono vittime civili, innocenti e predestinati, di guerre sanguinose o di lotte fratricide, o ancora sono privati dell'affetto e dell'amore dei loro genitori. Tutti noi conosciamo l'importanza fondamentale per un armonico sviluppo del bambino di due pilastri su cui poggia il futuro stesso dei nostri figli: la famiglia e la scuola. Se il bambino vive bene e sente l'amore e l'affetto della famiglia in cui vive e nel contempo è ben inserito nel contesto scolastico, ben accettato e opportunamente motivato, cresce forte nell'animo e maturo nella mente. L'asse portante scuola-famiglia deve lavorare in sinergia anche per riconoscere i primi segnali di difficoltà, insofferenza e richiesta di aiuto, a volte silenti e poco comunicati per timore o vergogna. Ecco l'importanza, tra le tante iniziative di diversi soggetti che si occupano e sostengono l'universo infanzia, della presenza di un riferimento continuativo e sempre presente: il Telefono azzurro che, nato con la nato con la finalità di difendere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rappresenta, con il suo numero telefonico 114, una vera e propria ancora di salvezza per i bambini in difficoltà o vittime di maltrattamenti e violenza.

un disegno di legge, semplice nella sua attuazione, che prevede l'obbligo di esposizione in tutte le pubbliche amministrazioni, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di cura, negli studi dei medici di base e dei pediatri di libera scelta di un cartello indicante il numero 114 Emergenza infanzia. Diffondere o conoscere chi può rispondere a una richiesta di aiuto può salvare spesso una vita. L'obiettivo deve essere sempre e comunque la tutela dei minori e dei più deboli: essere bambini è un diritto; per noi adulti è un dovere difenderli. *(Applausi)*. Signor Presidente, intervengo nell'Assemblea del Senato sul caso della consigliera comunale Giannino, che è stata oggetto grazie a tutti

mafiosa e vi fu in ballo anche una commissione di accesso agli atti da parte della prefettura di Roma. Chiedo allora nell'Aula del Senato, uno dei luoghi più solenni della nostra Repubblica, che le istituzioni non soggiacciano ad alcun timore e non si facciano prendere da nessuna reverenza. Chiedo che, dalla Commissione antimafia, alla prefettura, a tutte le istituzioni, venga acceso un faro sulla vicenda della un faro sulla vicenda della consigliera Giannino di Anzio e di un territorio che appare molto permeato di infiltrazioni e non solo. Chiedo quindi che tutte le istituzioni possano portare la loro solidarietà, ma soprattutto fare azioni concrete perché un gesto così vile non rimanga inascoltato in questa Repubblica. *(Applausi)*.

oggi è un giorno molto triste per la comunità e l'avvocatura nuorese, che piange la prematura scomparsa del nostro caro amico e collega, avvocato Salvatore Murru, uomo dal carattere mite e gentile, una persona seria e un grande professionista, già Presidente delle Camere penali di Nuoro. Egli lascia due ragazzi, Ignazio e Sebastiano, e una moglie, la mia collega Franca Paola, cui va il mio caloroso abbraccio. La città è assediata dalla malattia, il Covid. Non posso non ricordare le file di ambulanze fuori dall'ospedale San Francesco di Nuoro e il reparto Covid, con 33 pazienti e soli 6 medici. Come avvocato e rappresentante delle istituzioni in Senato, sono vicina a tutti i miei cittadini e a tutti i sardi e resto a loro disposizione nella lotta contro questa terribile malattia. Riposa in pace, Salvatore, sei stato e sarai sempre un esempio per tutti noi. Ringrazio l'Assemblea.

svolgo questo intervento per sollecitare la risposta a due interrogazioni. Già alcuni mesi fa una prima interrogazione è stata posta al Ministero della salute per chiedere di riprendere in mano una serie di passaggi chiave della legge n. 3 del che non prevedono l'uso del tabacco riscaldato e per riprendere in considerazione il danno alla salute che esso procura. Mi risulta che dall'Istituto superiore di sanità sia partita una documentazione, espressamente richiesta dal Ministero della salute, nella quale si affermava in modo chiaro e contundente che il tabacco riscaldato nuoce gravemente alla salute. Poi ho presentato una seconda interrogazione al Ministro dell'economia per chiedere per quale ragione una sostanza che oggettivamente nuoce gravemente alla salute dovesse godere di uno sconto fiscale pari al 75 in un momento in cui, com'è noto, in un'ottica di revisione e rivalutazione delle politiche fiscali, da una parte, si dichiara lotta all'evasione fiscale e, dall'altra, giustamente si cerca di andare incontro alle persone fin troppo tartassate da quello che possiamo chiamare il peso delle tasse.

il MoVimento 5 Stelle, attraverso la Casaleggio associati, abbia ricevuto dalla più importante azienda produttrice di tabacco riscaldato possiamo definire sovvenzioni, risorse economiche o finanziamenti, in misura decisamente consistente. A questo punto, il dubbio

pari al 75 per cento. Credo che ci siano tutte le premesse, compreso lo scandalo pubblico, per ottenere risposta a queste interrogazioni.